L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

come purtroppo già sapete, ieri a Casteldaccia, in provincia di Palermo, si è consumata l'ennesima tragedia sul posto di lavoro.

ci sono stati altri episodi, solo per citare gli ultimi, a Suviana, a Firenze, a Brandizzo, a Gioia del Colle e purtroppo potremmo andare avanti con una sfilza di luoghi. Mentre parliamo, stiamo attenti che già non arrivi un'altra drammatica notizia. Negli ultimi anni certamente sono aumentate le norme

e continueranno ad aumentare. Tuttavia, ci troviamo ancora a piangere delle vite spezzate, il che comporta la necessità di fare qualcosa tutti insieme, di fare uno sforzo straordinario perché questo tema sia una priorità per le Camere, per il Governo, per la società. Credo che ci sia bisogno abbiamo già detto non è più rinviabile - di un impegno di tutti, anche delle aziende e di coloro che sono preposti al controllo, persino degli stessi operatori, ai quali mi rivolgo perché non trascurino di esercitare essi stessi un controllo, una verifica, un'attenzione ancora maggiore. Questa ennesima tragedia sul lavoro, come ha detto il presidente Mattarella, deve riproporre con forza la necessità di una risposta comune.

la chiarezza non riporta in vita chi è morto. Certo, fa giustizia e quindi è auspicabile e auspicata, ma non possiamo accontentarci ogni volta di chiedere che si capiscano le ragioni, le responsabilità, le colpe di un dramma: occorre qualcosa di più, lo ribadisco, e non è la prima volta che da quest'Aula

Rivolgo veramente le nostre sentite condoglianze alle famiglie delle vittime, del ferito, a tutti gli altri soggetti, alle aziende e a tutti i Comuni coinvolti.

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 30 aprile scorso, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 16 maggio. Nella seduta di oggi saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Domani avrà inizio la discussione generale del disegno di legge costituzionale in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 8 maggio. La seduta di giovedì 9 maggio, con inizio alle ore 15, prevede il *question time* con la presenza dei Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e per le riforme istituzionali. Vi prego di prestare attenzione al fatto che nella mattinata di giovedì, alle ore 11, si terrà in Aula una cerimonia commemorativa delle vittime del terrorismo, con la presenza del Presidente della Repubblica. Tale cerimonia si svolge un anno alla Camera e un anno al Senato. Quest'anno avremo qui il Presidente della Repubblica. Il calendario della prossima settimana prevede il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. Mercoledì 15 maggio, a partire dalle ore 15 e senza orario di chiusura, sarà discusso il decreto-legge in materia di agevolazioni fiscali, anche ove non concluso in Commissione, con eventuale seguito nella giornata di giovedì 16. maggio, alle ore 15, avrà luogo il *question time.* Martedì 14 maggio, in apertura di seduta, sarà commemorata la figura dell'ex senatore Nino Diremo in seguito se, come è possibile, nel corso dei prossimi lavori sarà prevista anche una votazione per l'elezione

Signor Presidente, come è noto, il calendario dell'Aula non è stato votato all'unanimità nella Conferenza dei Capigruppo; in particolare c'è stata la contrarietà di diversi Gruppi di opposizione. dovuto ad un'accelerazione e a un calendario che riteniamo di non dover accettare rispetto alla riforma costituzionale sul premierato, che porta, ad esempio, alla situazione quasi surreale di avere la scadenza degli emendamenti che coincide con l'inizio della discussione generale. È evidente che una discussione su una riforma così importante, che si può condividere o meno, ma che rimane di enorme

Adesso non entro nel merito della riforma proposta dal Governo e dalla maggioranza, che modifica in modo a nostro avviso pericoloso i pesi e i contrappesi del dettato costituzionale, ma ritengo che quest'Assemblea non abbia nessuna urgenza di comprimere i tempi del dibattito. La nostra proposta è duplice

alla discussione di una mozione che abbia ad oggetto il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in modo da poter condividere tra tutte le forze politiche qualche proposta

nella giornata di giovedì, di una mozione possibilmente unitaria sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, rimandando di due settimane l'inizio della discussione generale sul disegno di legge di riforma della Costituzione, con l'introduzione di un *unicum*

mi limito a sostenere la proposta del presidente Patuanelli e ad integrarla eventualmente con ulteriori provvedimenti, perché condividiamo con il presidente Patuanelli la richiesta di uno slittamento dell'inizio della discussione generale sulla riforma costituzionale e di integrazione del calendario - così come ci eravamo detti in Conferenza dei Capigruppo con alcuni provvedimenti che possono essere inseriti. Ci sono delle mozioni che i Gruppi parlamentari hanno segnalato e purtroppo, anche riallacciandoci all'apertura della seduta da lei fatta, il Gruppo Partito Democratico ha chiesto

questione del lavoro forse è bene che avvenga in un clima di maggiore coesione generale. Comunque con altre mozioni, diciamo così.

Signor Presidente, abbiamo espresso già in sede di Conferenza dei Capigruppo con le altre forze dell'opposizione, come lei ha ascoltato in quella sede e come naturalmente avrà capito anche adesso e come anche i colleghi stanno comprendendo in questi minuti, le ragioni per cui abbiamo espresso un dissenso rispetto alla scelta che è stata fatta e che sarà da qui a pochi minuti imposta a quest'Assemblea con un voto: il modo davvero peggiore per cominciare l'*iter* di una riforma costituzionale.

l'assetto istituzionale del Paese e la sua architettura istituzionale. Anche in mancanza di una condivisione di merito, sarebbe particolarmente utile almeno mettersi d'accordo sul percorso. Poi si vede se anche sul merito ci sono elementi di condivisione o meno, e in questo caso, almeno stando a quanto accaduto in Commissione nel corso di questi mesi, evidentemente ci sono posizioni diverse. Devo dire che pensavo e continuo a pensare che almeno sul metodo, cioè sul

che trovo davvero molto grave che si voglia fare questa forzatura. Perché la si vuole fare? Qual è il motivo per cui l'Assemblea del Senato deve cominciare a discutere la riforma costituzionale adesso? Stiamo forse parlando di un decreto-legge che scade, signor Presidente? Abbiamo una scadenza prevista dalla legge, per cui da qui a qualche settimana, venuta meno la scadenza, viene meno il decreto? Oppure parliamo di un provvedimento di altra natura, ossia di una riforma costituzionale che peraltro, come sappiamo, necessita di un doppio passaggio parlamentare, ossia di due passaggi alla Camera e due passaggi al Senato? Erano stati molto saggi i Padri costituenti all'epoca quando previdero questo tipo di andamento, perché evidentemente immaginavano che la riforma costituzionale

c'entra forse qualcosa questa anticipazione che si vuole fare e questo voto che probabilmente si vuole dare nelle prossime settimane

anche appreso - non lo sapevo, perché pensavo che Giorgia fosse il nome di battesimo della Presidente del Consiglio - che invece è anche una sorta di soprannome. Ho scoperto, signor Presidente, che alle elezioni europee che verranno

quando c'è scritto "detto" sul nome di un candidato è perché evidentemente il nome del candidato è diverso dal nome che si scrive. Invece in questo caso, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, scopriamo che ci si può candidare alle elezioni con il proprio nome e ci si fa dire "detto" sempre con il proprio nome, non con un nome diverso dal proprio. I manifesti di Giorgia sono dappertutto nel nostro Paese e contemporaneamente si forza sulla necessità di votare in prima istanza il premierato, prima delle elezioni europee. Ma pensate davvero che qualcuno non capisca? Davvero pensate che c'è qualcuno che possa non avere la minima percezione di quello che sta accadendo non pensare che state piegando la riforma costituzionale a un interesse di parte e di propaganda? Lo state facendo, evidentemente

Lo vedo tutti i giorni, lo vedo il 25 aprile, quando si fa fatica a riconoscere, per esempio, la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana. Quindi, capisco bene che ci possa essere qualche elemento di allergia nei confronti della Costituzione; lo capisco, del resto è una cosa nota che sappiamo da molti anni e da molti decenni. Questo evidentemente non mi sorprende. Tuttavia penso, signori Ministri, che siccome su quella Costituzione giurate, giurate, nei confronti di quella Costituzione dovreste mostrare il rispetto che merita e dovreste perlomeno evitare di piegare il cambiamento della Costituzione a un interesse di parte facendolo nel modo che state scegliendo, perlappunto con una forzatura, subito prima delle elezioni europee, con manifesti che coprono tutte le strade e tutte le piazze delle nostre città, che di fatto stanno facendo immaginare una sorta di premierato anticipato. Davvero voi pensate che si possa fare tutto? Guardate che avere la maggioranza dei voti, aver vinto le elezioni politiche, cosa che - com'è evidente tutti vi riconoscono, perché naturalmente sta nei numeri, non vi autorizza ad immaginare di stravolgere in questo modo le regole di fondo. Le regole prescindono dai numeri; i numeri determinano le maggioranze e le minoranze, poi però ci sono le regole che dovrebbero impegnare tutti, maggioranze e minoranze. Allora, credo francamente che il voler fare questa forzatura adesso e voler portare a casa questo scalpo, perché di questo si tratta, evidentemente ha delle ragioni che non c'entrano niente con la necessità di fare un approfondimento serio su una riforma - non la raccontate in maniera diversa da quella che è che non è vero che tocca leggermente i poteri di questa Costituzione, ma cambia radicalmente la Costituzione di questo Paese *(Applausi)*, mettendo in discussione radicalmente quell'idea di Governo parlamentare su cui si è fondata la Repubblica italiana per decenni, mettendo clamorosamente in discussione quell'equilibrio dei poteri che dovrebbe essere sempre la prima regola attorno alla quale si definisce una democrazia. Poi, naturalmente, entreremo nel merito già domani mattina, quando presenteremo le pregiudiziali, ma voglio stare al metodo adesso e voglio sapere qual era la ragione di forzare. Perché dovete portare questo scalpo? Lo dovete fare probabilmente perché alla Camera è in discussione il disegno di legge sull'autonomia differenziata ed evidentemente i due partiti principali che compongono l'alleanza di Governo avevano bisogno di questo scambio reciproco? Perché nel momento in cui si fa l'autonomia alla Camera, bisognava necessariamente fare anche il premierato al Senato? Evidentemente le ragioni sono queste, non hanno nulla a che fare con una normale dialettica democratica. Qui non si sta chiedendo di essere tutti d'accordo. Si può essere contrari, naturalmente, e si può avere anche un dissenso, com'è evidente, su come e se cambiare la Costituzione. Io, per esempio,

nel merito di nessun intervento, però voglio rassicurare lei e tutta l'Assemblea che il rispetto delle regole è garantito da me, dal Consiglio di Presidenza e dalla riunione dei Capigruppo. Ci possono essere divergenze sul percorso, e ci sono, ma non vi è nessuna violazione di regole, anzi, nel caso specifico devo dire

circa 90 iscritti a parlare in discussione generale, oltre alle pregiudiziali. Non mi pare che ci sia una violazione di regole. Va benissimo tutto, ma vi prego di non dire che c'è una violazione di regole, perché attiene alla mia responsabilità

ribadire un antico distico che chi ha iniziato a fare politica qualche anno fa si sentiva ripetere quasi in maniera da giaculatoria di chiesa, e cioè che in politica la forma è sempre sostanza. la discussione sulla forma con la quale l'Assemblea si appresta ad affrontare e licenziare un provvedimento così importante non è né una vicenda oziosa, né una questione leziosa. È una questione strutturale e lo è, signor Presidente, ancor più a fronte del modo con il quale la Presidenza ha ritenuto di dovere investire la Conferenza dei Capigruppo dell'organizzazione di questi lavori. Infatti, e lo dico senza amor di polemica, ma per cercare di portare un contributo che vada nella direzione di sgombrare il campo rispetto all'introduzione di spurie modalità di interpretazione di questa nostra odierna attività, la proposta che ha fatto la Presidenza in seno alla Conferenza dei Capigruppo è stata eccessivamente zelante,

la proposta con la quale la Presidenza ha impostato questi nostri lavori è sembrata quasi interpretare l'esame del provvedimento alla stregua di una ratifica alla quale quest'Assemblea è per troppe volte stata chiamata, come se la riforma costituzionale fosse la traduzione in legge di un decreto che, una volta conclusa

discussione di un procedimento una volta che sia concluso l'esame in Commissione. Su questo noi diamo atto che la Presidenza si sta muovendo nel rango delle prerogative e dei doveri che possiede. Si è concluso in Commissione un *iter* ed è giusto doveroso che l'Assemblea inizi la discussione. Il punto, però, è la modalità con la quale questa discussione si apre, apre, immaginando di poter aprire e chiudere la discussione in un arco temporale già predefinito, come era nei desiderata originali. Solo a seguito degli interventi in sede di Conferenza dei Capigruppo questo arco temporale, già circoscritto e predeterminato, è limitato all'interno del mese di maggio, come se l'esame del provvedimento di riforma della Costituzione fosse l'approvazione di un decreto. è evidentemente una questione che tradisce il retro pensiero circa il fatto che l'Aula debba sostanzialmente e fattualmente ratificare l'operato della Commissione. *(Applausi)*. Così non è: questo il primo punto, colleghi. È doveroso che l'Aula inizi la discussione, ma è altrettanto doveroso che la discussione si sviluppi in tempi e modalità consoni alla possibilità di entrare nel merito delle proposte emendative,

Dico ciò riprendendo un precedente, signor Presidente, che mi sono andato a studiare e che forse potrebbe essere utile per l'impostazione dei nostri lavori. Un'analoga situazione si verificò nella XVII legislatura, quando il Governo presentò

Il Senato iniziò la discussione il 9 luglio 2014 e concluse le votazioni l'8 agosto del 2014. Vi furono interventi sull'andamento dei lavori, 163 interventi in discussione generale, che, nettizzandoli rispetto alla riduzione del numero dei parlamentari, corrisponderebbero a 108 parlamentari senatori che potrebbero intervenire nell'ambito della discussione generale. Vi furono 26 sedute, 744 interventi sugli articoli con relative votazioni, 144 ore di discussione. Questo è il *range* di una discussione parlamentare di modifica costituzionale almeno pari a quello di cui stiamo discutendo. Io credo sarebbe stata buona cosa se, partendo dai precedenti, si fosse immaginato di investire il nostro lavoro circoscrivendo, all'interno di un perimetro di questa natura, una ipotesi dei nostri lavori. Invece, ci siamo trovati nella condizione per la quale dapprima si pensava di chiudere

europee. Questo sarebbe un errore, contro l'interesse stesso dei proponenti della riforma, perché significherebbe introdurre nel dibattito elementi spuri che nulla hanno a che vedere con le questioni di merito. Dividiamoci pure sui palchi dei comizi delle elezioni europee; ma, quando ci troviamo a discutere della Costituzione, facciamo lo sforzo di trovare un minimo comune denominatore. Se traduciamo gli elementi della divisione partitica nella costruzione degli elementi strutturali della nostra democrazia, infatti, noi non rendiamo un buon servizio alla qualità del nostro lavoro. E vorrei anche dire, ai colleghi della maggioranza, che neppure voi rendete un buon servizio al vostro lavoro, perché rischiate di introdurre, all'interno di questi lavori, elementi di perturbazione che inevitabilmente emergerebbero nel corso d'opera dei nostri lavori. immaginiamo di poter impostare i lavori nei termini che ho detto, attraverso l'impiego temporale cui ho fatto riferimento, magari ipotizzando di dilatare il termine della presentazione degli emendamenti, che è fissato per domani mattina alle 10. Siccome sappiamo tutti, cari colleghi, che la prima lettura del Senato è l'unico momento nel quale potremo realmente intervenire in modo modificatorio modo modificatorio perché, dopo che si sarà andati in seconda lettura alla Camera - e quella sarà la reale occasione nella quale, anche per motivi di merito su cui non entro, si modificherà il testo - noi qui dovremo correre con gli stivali delle sette leghe senza poter cambiare assolutamente nulla, avendo qualcuno già detto che tanto l'obiettivo finale è il *referendum*. Siccome noi crediamo ancora, anzi crediamo fermamente che la funzione del Parlamento, soprattutto nel momento in cui viene trasformato in Assemblea costituente, non è né di ratifica né di carattere propagandistico; e siccome noi abbiamo delle opinioni di merito - domani saranno espresse anche sulle questioni pregiudiziali dalla collega Musolino - che per alcuni aspetti ci differenziano dalle altre opposizioni, a maggior ragione perché abbiamo questa posizione riteniamo che lo strumento di garanzia di tutte le opposizioni per entrare nel merito della possibilità di articolare al meglio le proprie posizioni sia un elemento che debba essere tenuto in assoluta considerazione anzitutto dalla maggioranza.

ma non è previsto per quella data il voto conclusivo, per cui si potrà andare avanti se ci saranno

non perché speri di far cambiare idea alla maggioranza, perché naturalmente andrà avanti come ha sempre fatto, sorda e cieca, ma perché

come è stato ricordato anche poco fa dal collega Enrico Borghi - in realtà un termine è stato messo ed era quello del 21 maggio; poi, di fronte alle proteste dell'opposizione in sede di Conferenza dei Capigruppo, questo limite temporale è diventato improvvisamente più sfumato, ma il gioco è chiarissimo. Al di là di questo, la mia è una denuncia - e quindi non è per i colleghi di maggioranza, che sono certa, purtroppo, non ascolteranno - per chi potrà ascoltare al di fuori di questi palazzi. riforma costituzionale nasce già non condivisa, nasce già da una finta volontà di ascolto e condivisione: era già tutto predeterminato. alle delegazioni che sono andate dalla ministra Alberti Casellati e poi da Giorgia. A questo punto, credo di potermi prendere la libertà di chiamare il Presidente del Consiglio Giorgia, visto che lo fa scrivere addirittura sulle urne. PRESIDENTE. È il suo nome. Siamo andati anche da Giorgia, ma naturalmente l'ascolto era finto, perché avevate già in mente come intervenire, stravolgendo la nostra Costituzione. Vi siete Vi siete vantati che questa è una riforma chirurgica e non invasiva; chirurgica come un taglio netto alla giugulare della nostra Costituzione, perché questo è quello che questa riforma fa: dissangua la Costituzione repubblicana e la trasforma in qualcos'altro, qualcosa di lontanissimo da ciò che i nostri Padri e Madri costituenti avevano immaginato e voluto per il nostro Paese. E lo fate E lo fate in maniera assolutamente non condivisa e con la forza dei numeri. Devo citare nuovamente il collega Borghi, perché ha fatto alla famosa riforma Renzi del 2014 quasi come ad una buona prassi, perché non so quanti interventi e quante ore di discussione Eppure, anche per quella riforma non si cercò una condivisione trasversale, ma si andò avanti con la forza dei numeri. conto, colleghe e colleghi, che le riforme costituzionali che vengono imposte con la forza dei numeri non portano bene a chi le impone. Quindi state in guardia rispetto a quello che fate, perché il popolo italiano non si fa prendere in giro così facilmente. Anche oggi, con il voto del calendario, potrete imporre l'inizio della discussione di questa riforma già a partire da domani e magari anche vederla approvata secondo i desideri di Giorgia, prima dell'inizio della campagna elettorale per le europee. È questo quello che volete: portare lo scalpo del Sud Italia alla Lega Nord con l'autonomia differenziata e lo scalpo della Costituzione repubblicana a a quelli che sono i vostri elettori, che state ingannando comunque con degli *slogan* fasulli. *(Applausi)*. Noi non possiamo far altro che opporci con la forza della ragione: i numeri non sono dalla nostra parte, ma vi chiediamo di aspettare perlomeno questo tempo, in modo da non strumentalizzare una riforma costituzionale di tale peso e di tale importanza per il Paese e di iniziare la discussione dopo che il Paese si sarà espresso per il Parlamento europeo.

Ricordo che può intervenire un senatore per Gruppo, ma per il Gruppo Misto mi arrogo il diritto di dare la metà del tempo, tre minuti, anche alla senatrice Signor Presidente, penso sia emerso anche durante i lavori in Commissione affari costituzionali che Azione non ha un atteggiamento ostruzionistico nei confronti della riforma costituzionale. Noi abbiamo avanzato un modello diverso, che è il modello tedesco. Siamo critici, ma riconosciamo il diritto della maggioranza di procedere alla riforma costituzionale. Vengo a quello che però non ci convince, signor Prima il collega Borghi diceva che la forma è sostanza. Io aggiungo che anche la scelta di tempo in politica è un fatto non secondario. secondario. Poiché dobbiamo ammettere tutti che questo non è un mese come gli altri, ma è il mese nel quale le forze politiche si confrontano e spesso si scontrano di una campagna elettorale plurima che riguarda le europee, ma anche le elezioni amministrative; e poiché questo Paese non ha trovato una via produttiva alle riforme costituzionali, perché sia la via dell'articolo 138 della Costituzione che la via della bicamerale sono fallite entrambe, penso che quello che non dobbiamo fare sia ripercorrere gli errori del passato.

ma sostanzialmente una profonda conflittualità sull'andare a votare il provvedimento, sull'esaminarlo o meno. Io credo che il buonsenso e la saggezza suggeriscano un supplemento di riflessione. Presidente, nel frattempo, anche chi ha votato, come la sottoscritta, a favore dell'autonomia differenziata, non può non considerare che i LEP non sono stati ancora minimamente finanziati. Non c'è un passo avanti sui LEP. Credo allora che, per evitare polemiche e contrapposizioni; per dare la sensazione di un intendimento vero a realizzare le riforme, dovreste cominciare a dare continuità al finanziamento dei LEP dentro l'autonomia differenziata che quest'Aula ha già analizzato; far passare la campagna elettorale e, poi, provare a trovare una via condivisa per costruire riforme costituzionali che non siano accomunate dallo stesso destino di quelle precedenti di altri Governi che, essendo frutto di una posizione solo di maggioranza, anche quando erano riforme organiche, alla fine si sono schiantate contro un muro. Affrontare un tema come la riforma costituzionale in piena...

quindi prescindendo al momento dal merito, da quello che sentiamo e ascoltiamo, io voglio innanzitutto rilevare che noi arriviamo a questa discussione mesi dopo le elezioni. La tematica dell'elezione del Presidente della Repubblica non si è più fatta; quella del *Premier* è già un modo per andare incontro a delle tesi diverse, dal momento che c'erano varie declinazioni del principio di democrazia diretta. Io, per esempio, personalmente sarei favorevole, come tanti, a un presidenzialismo ancora diverso. L'elezione del *Premier* però è già stata concepita dalla maggioranza come un'apertura

sul calendario, non nel merito, dopo mesi di confronto in Commissione, dove non mi risulta sia stato coartato nessuno. Il dibattito c'è stato, sono stati presentati emendamenti, proposte e modifiche. Lo stesso Governo e la maggioranza hanno modificato il testo in corso d'opera. E, siccome questa procedura prevede la doppia lettura - come è giusto che sia - del Senato e della Camera per una modifica della Costituzione, io immagino che anche nel dibattito e nel confronto d'Aula al Senato ci saranno delle modifiche ulteriori. Leggo vari approcci: c'è chi non condivide l'aver tolto dalla Costituzione la soglia di sbarramento delle cifre riguardanti la legge elettorale. Io invece ho ritenuto giusto

penso a Ceccanti ed altri - hanno fatto delle altre proposte che discuteremo e prenderanno forma di emendamenti. La cosa non mi scandalizza. Anche nella maggioranza ci sono delle voci che hanno espresso

Siamo in ritardo con gli italiani con i quali ci siamo impegnati a fare una riforma di questo genere. Non siamo in anticipo soffocatorio del dibattito parlamentare. Ma, per carità. Poi, entrando nel dettaglio,

nel provvedimento. A volte si mette nel calendario la data di votazione, alcune settimane dopo. Qui non è stato nemmeno indicato se il 21 maggio ci sarà una si vedrà. Se ci sarà una discussione generale, sarà molto ampia, e vi parteciperanno tutti i colleghi che vorranno ed è già previsto. Si è ipotizzato che domani inizi una discussione

una fretta spasmodica è una cosa infondata e non vera, rispetto ai tempi della storia e ai tempi della cronaca. Questa è la realtà dei fatti, cari colleghi. Inoltre - questo lo diremo anche domani, quando ci saranno le pregiudiziali di merito - noi non siamo in anticipo di un paio di settimane: siamo semmai in ritardo di trent'anni rispetto a una riforma materiale della Costituzione che l'elettorato ha già fatto. *(Applausi).* Caro collega Boccia, allarga le braccia quanto vuoi. Giorni fa sono stato invitato da Franco Bassanini - penso a sinistra sia conosciuto - a un seminario del suo centro studi

che, quando votano, o vince Prodi, o vince Berlusconi, o vince la Meloni, o vince non so chi era il candidato dall'altro lato, o vince Veltroni. Gli elettori dal 1994 votano pensando di scegliere chi guida il Governo. È la Costituzione che è in ritardo sulla democrazia reale che il popolo italiano vive dal 1994. *(Applausi)*. E ne avete fruito anche voi, quando avete vinto. Questa è la realtà. Quindi siamo in anticipo di una settimana? Ci dovrebbero fischiare i nostri elettori, quelli del centrodestra: siamo in ritardo di trent'anni rispetto a un'interpretazione legittima, democratica, popolare della scelta dei Governi. ci sono state - ma lì si dovrebbe discutere delle leggi elettorali - legislature in cui non c'erano maggioranze e in cui poi finiva sempre uno del Partito Democratico a fare il Presidente del Consiglio, quando non c'erano le maggioranze. *(Applausi)*. i Governi Letta, Gentiloni o altri Governi. È chiaro che a voi non piace questo sistema, perché volete pescare nel torbido del sistema indifferenziato, dove non si sa chi vince. Allora accettate questa discussione sulla democrazia del Paese, che viene rafforzata dal premierato lasciamo perdere il presidenzialismo. Poi domani sulle pregiudiziali parleremo anche dei poteri. Una volta il Presidente del Senato è stato criticato perché avrebbe criticato i poteri del Presidente della Repubblica. Io ho capito cosa voleva dire il presidente La Russa, che poi lo ha spiegato: a volte le carenze del sistema attuale hanno costretto, per bene di Patria, i Presidenti della Repubblica a un'azione suppletiva: scegliere i Governi quando non c'erano maggioranze definite, perché il Paese doveva essere governato. È successo questo in Italia. La constatazione è che semmai i poteri dei Presidenti della Repubblica si sono allargati, forse per difetto del sistema politico, che non era bipolare e aveva tre o per circostanze che hanno anzi consentito a quei Presidenti di garantire la continuità della Repubblica e della nostra democrazia. Semmai è un merito, ma è un dato di fatto che quei poteri si siano allargati. In quella lezione di diritto costituzionale materiale ho raccontato alcuni episodi. Volete sapere come si eleggono i Vice Presidenti del CSM? Volete sapere i Presidenti della Repubblica come si occupano di queste vicende? Lo racconteremo in costanza di dibattito. E non mi scandalizzano queste cose, cari colleghi. Non mi scandalizzano, perché poi qualcuno deve - come dire - aiutare la democrazia ad esprimersi, quando noi non riusciamo a eleggere i giudici della Corte costituzionale o in altre situazioni. Io credo che non ci sia alcuna fretta del Regolamento. La proposta che è uscita a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo consente di discutere nel mese di maggio, e forse non discuteremo. C'è poi la storia secondo cui "devono votare prima delle elezioni europee". Ma, se siamo in ritardo di trent'anni, io non sono preoccupato, avendoli vissuti questi anni in Parlamento, se si voterà il 28 maggio o il 18 giugno, rispetto a un appuntamento con la storia. Ci sarà poi la lettura della Camera e poi il provvedimento tornerà al Senato: quanta acqua deve scorrere sotto i ponti del Tevere prima che questa riforma prenda corpo secondo le regole costituzionali!

è la realtà, che è perfettamente compatibile con la democrazia repubblicana, con la democrazia americana, con la democrazia francese, con tutte le democrazie che in vario modo danno più potere ai cittadini nella scelta.

attuare uno degli aspetti del suo programma, un dibattito che dura da decenni e che nella coscienza democratica - parlate con i vostri elettori - è già in vigore, secondo molti. Credo che la discussione di merito avverrà e parleremo dell'emendamento, del subemendamento e quant'altro; poi verranno le leggi elettorali e verrà altro. Signor Presidente, noi rivendichiamo il diritto di attuare quella proposta di calendario uscita a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo. Non siamo a strangolare le settimane di dibattito. Siamo semmai - e mi scuso con i nostri elettori - in ritardo di qualche anno e vorremmo finalmente una democrazia che decida su se stessa.

La notizia che il presidente Gasparri ha appena dato all'Assemblea è che parteciperanno alla discussione. Purtroppo in questi mesi, presidente Gasparri, abbiamo cercato di

Lei sa che, se c'è un tema particolarmente caro a me, al presidente Patuanelli, al presidente De Cristofaro, alla presidente Unterberger, al collega la tutela spasmodica della credibilità di quest'Assemblea e, quindi, del Parlamento. Ogni volta ci mettiamo nella condizione di difendere fino in fondo le prerogative del Parlamento. Signor presidente Gasparri, lei

perché semplicemente siete stati assenti, siete stati silenti, siete stati supini, siete stati obbedienti. La cosa che ci preoccupa, signor Presidente, e che dovrebbe preoccupare tutti in quest'Aula è che lo avete fatto perché una riforma costituzionale come questa, che è su su proposta del Governo, è un ordine per uno scambio politico tra i due principali partiti di maggioranza. All'improvviso vi svegliate perché di là, a Montecitorio, parte il miglio finale sull'autonomia che spacca l'Italia e che abbiamo denunciato qui più volte.

non rendere solvibile, liquido questo scambio, sulla pelle delle italiane e degli italiani. La democrazia, signor presidente La Russa, è sempre un esperimento: non è data, non è una certezza; è un esperimento che non finisce mai e che viene rafforzato o indebolito dalle classi dirigenti che ne hanno la responsabilità. Questa volta, per i numeri non per la politica, tocca a voi avere questa responsabilità. Guardate che la qualità della democrazia incide sulle libertà. Al presidente Gasparri, signor Presidente, vorrei ricordare - perché forse lo ha dimenticato nel suo intervento

di associazione, di diritto alla vita, di vita politica. Voi pensate che tutto questo non venga messo in discussione dall'impianto folle che avete messo su? Non se la prenda la ministra Casellati, che ha tentato di tenere insieme "pere e mele", ma questa è una riforma della nostra Costituzione che avviene per ordine del Governo di turno. Ce ne sono stati tanti, anche questo passerà

questo disegno di legge governativo, presentato in un modo, poi stravolto e cambiato completamente - tutti gli ex presidenti della Consulta e tutti i Presidenti emeriti di fatto vi hanno detto che con questa riforma non si va lontano, e tutti i costituzionalisti, tranne l'estensore della riforma, hanno detto che era un pasticcio e un disastro - non sentite sulle vostre spalle la responsabilità di quello che state facendo? Noi chiediamo lo slittamento perché intanto pensiamo che lo scambio vergognoso sul piano politico tra Lega e Fratelli d'Italia, che plasticamente si vede anche nelle due Aule, tra Senato e Camera, umili la Repubblica e vada fermato. Ma, se anche non volete fermarlo, provate ad entrare nel merito fino in fondo; assumetevi la responsabilità, colleghe e colleghi della maggioranza, di fare una proposta parlamentare da mettere sul tavolo del Governo di turno, del Governo *pro tempore*. Invece no: siete lì che guardate,

Nel dibattito in Commissione affari costituzionali affari costituzionali non abbiamo sentito tante proposte. Ne avremmo volute altre e non ce l'abbiamo fatta. Ma la cosa che vogliamo sottolinearvi oggi, prima del voto, è che far slittare di alcune settimane questo passaggio potrebbe consentirci di ritrovare le ragioni di modifiche che incidono pesantemente sulla funzione del Presidente della Repubblica e lo abbiamo denunciato più volte. Una volta poi costruito questo impianto e portato al voto, immaginiamo che - così com'è stato fatto in Commissione - anche in Aula la maggioranza non presenterà emendamenti o presenterà presenterà ordini del giorno connessi ad impegni possibili durante il dibattito nelle diverse letture. Signor Presidente, noi pensiamo che questa sia un'occasione che riguarda non un Gruppo parlamentare o un altro, ma la credibilità di tutto il Parlamento. Dietro ogni articolo della Costituzione - ricordava il presidente Pertini - ci sono centinaia di morti della Resistenza Resistenza *(Applausi)*, dietro ognuno dei 139 articoli. Sì, presidente Gasparri, probabilmente dovremmo leggerli qui in Aula tutti i 139 articoli per capire quanto è bella la nostra Costituzione. perché è scritta, perché è rigida, perché è lunga, perché laica, perché democratica, perché programmatica e perché soprattutto - signor presidente La Russa - è votata dal popolo. È lì che ritorniamo:

e gli italiani la ritengono la propria Costituzione *(Applausi)*. Allora, signor presidente La Russa, siccome per proposta e imposizione del Governo ci ritroviamo in questa condizione sia per la riforma della Carta fondamentale, da una parte, che per un'autonomia che spacca l'Italia, dall'altra, facciamo davvero l'ultimo appello prima del voto del calendario: fermatevi finché siete in tempo. Noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità democratiche per fermare questo scempio.

potuto evitare di intervenire. Sentendo però il collega del Partito Democratico continuare a insistere sulla questione legata allo scambio politico tra la Lega e Fratelli d'Italia sul tema dell'autonomia e del

*(Applausi)*, visto che sono mesi che parlate del campo largo che alla fine è diventato stretto e poi minato, per non dire altro. In una coalizione ci sta benissimo che ogni partito che ne fa parte, quando presenta un programma elettorale, un programma politico, metta in evidenza le proprie priorità.

la Lega voleva l'autonomia, Fratelli d'Italia puntava su una maggiore stabilità del Governo - presidenzialismo o premierato è una scelta che è stata fatta in un secondo momento - e Forza Italia voleva la riforma della giustizia. Cosa c'è di più trasparente e di più chiaro nel voler portare avanti tutte e tre le riforme nello stesso identico momento, per dare dimostrazione ai nostri elettori che non li vogliamo prendere in giro? Io posso capire che dall'altra parte si dica che non si è d'accordo. Ci sta: ognuno legittimamente la pensa alla propria maniera e utilizzerà tutti gli strumenti che la democrazia e i regolamenti gli mettono a disposizione per poter contrastare quello su cui non è d'accordo. Anzi, il confronto è bello

è assolutamente nella logica dell'equilibrio e del buonsenso che, come contrappeso, si diano più poteri ai territori. È un elemento talmente trasparente, semplice e se volete anche banale, che davvero fatichiamo a comprendere come quelli del Partito Democratico e delle opposizioni non riescano a capirlo. Davvero fatichiamo a comprenderlo. Nessuno scambio, massima trasparenza e massima volontà di portare avanti le riforme. Poi - come ha detto bene il collega Gasparri - non vi si chiede la settimana prossima di approvare la riforma. Ci sarà una discussione, ci sono gli emendamenti; avrete modo di poterli presentare, di votarli, di poter presentare dei miglioramenti al testo rispetto al lavoro che è stato fatto in Commissione. C'è un confronto politico in Aula che è più che legittimo.

chiedendo la calendarizzazione di questo provvedimento, così come è stato calendarizzato il provvedimento sull'autonomia differenziata, è che esso è una parte del programma elettorale sulla quale ci siamo impegnati davanti agli elettori. Gli elettori hanno liberamente scelto di dare fiducia alla coalizione che ha presentato questo programma e noi riteniamo che gli impegni presi con gli elettori siano impegni da mantenere.

Questo vorrebbe dire che noi, per tenere la stessa velocità, avremmo dovuto avere il voto finale in Aula, nell'Assemblea legislativa, il 14 marzo scorso. Quindi, come anche detto dal presidente Gasparri, semmai siamo in ritardo,

al *leader* del Partito Democratico, Elly Schlein, ha detto che, se c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, non c'è dialogo e impediranno in tutti i modi di andare avanti. È legittimo. L'ostruzionismo è una pratica pienamente legittima e fortemente radicata nei sistemi democratici. Sta di fatto, però, che non è cercare non è cercare il dialogo presentare 2.600 emendamenti, un migliaio dei quali sono stati dichiarati o inammissibili o preclusi per l'approvazione di altri emendamenti. Di conseguenza, ne sono stati esaminati

straordinaria proliferazione di micromodifiche, e con microdifferenze tra un emendamento e l'altro. se non c'è stato questo dialogo, che noi pure auspichiamo, non è da attribuirsi alla maggioranza, ma alle cose che l'opposizione ha dichiarato e ha coerentemente messo in atto.

Tornando alla riforma di ormai dieci anni fa, promossa da un Governo guidato da un Presidente del Consiglio che era il *leader* del Partito Democratico e che oggi è presente in un altro Gruppo, ma comunque qui autorevolmente rappresentato, non di persona (perché oggi non c'è), ma dal presidente del suo Gruppo Enrico Borghi, ricordo un emendamento premissivo all'articolo 1 per evitare di dover fare troppi voti e per precluderne molti altri in Aula. Pertanto, anche in quel caso non abbiamo molto da imparare; semmai, potremmo avere la tentazione di imitare questo modo di limitare - in questo caso, davvero - la discussione. Come dicevo, dall'anno scorso abbiamo fatto 76 sedute in Commissione,

di sacralità e di rispetto verso la Costituzione, quella Costituzione che è costata grandi sacrifici di tanti; era sempre quella però la Carta della quale voi volevate cambiare 53 articoli: allora a quell'epoca non era sacra la Costituzione? Non c'era più bisogno di rispettarla? Ricordo anche che la riforma dell'autonomia differenziata che oggi affrontiamo con un disegno di legge applicativo è stata voluta dal centrosinistra, con una maggioranza di ben quattro deputati nella Camera da 630 componenti, nell'anno 2000. Era sempre quella la Costituzione che avete cambiato e che adesso dite che verrebbe stravolta. L'autonomia differenziata è stata votata dalla maggioranza di centrosinistra nell'anno 2000, per cui anche in quel caso la Costituzione era sempre la stessa, quella che dobbiamo guardare giustamente con rispetto. Noi sosteniamo che la Costituzione va guardata con rispetto non soltanto a parole, ma va rispettata e non va interpretata secondo nuove concezioni. La Costituzione è tutti coloro che hanno combattuto e che hanno lavorato hanno voluto scrivere quella Costituzione e non quella che oggi qualcuno può pensare di interpretare, cioè di stravolgere, il che è molto peggio. Se si vuole cambiare la Costituzione, si propongono modifiche, specialmente nella prima parte. Non si può andare avanti a forza Pertanto noi auspichiamo che in quest'Aula si possa procedere con l'esame di questa riforma a attribuiamo grande importanza. Io credo che tutti coloro che si oppongono (naturalmente più che legittimamente) a questa riforma dovranno spiegare ai cittadini italiani perché non vogliono che siano i cittadini stessi, attraverso il loro voto, a scegliere chi governa e che invece dobbiamo continuare ad avere Governi guidati da chi non è mai stato eletto da nessuno. Anche in questo quella riforma non era stato eletto da nessuno, se non dai rispettabilissimi cittadini di Firenze, che però non sono il popolo italiano e che lo avevano eletto sindaco e non capo del Governo italiano. Noi, invece, vorremmo essere simili a quello che succede in altri Paesi, dove non cambia un Esecutivo all'anno, dove c'è stabilità dei Governi e vorremmo farlo con strumenti appropriati che vadano nel solco della nostra tradizione costituzionale, che è anch'essa diversa da quelli degli altri Paesi.

Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 92 del nostro Regolamento, desidero portare all'attenzione di quest'Assemblea un tema che ci ha visti anche protagonisti in passato, ma che ora diventa assolutamente dirimente e fondamentale. Mi riferisco al caos che si è venuto a creare sulla questione delle concessioni balneari.

su chi è favorevole alle gare, su chi vorrebbe prorogare, su chi invece le gare non le vorrebbe mai fare, perché non è questo il punto della questione. alla vigilia dell'apertura della stagione ci sono più sentenze che tra l'altro finiscono anche per contraddirsi, abbiamo visto la recente sentenza del Consiglio di Stato dire fondamentalmente che bisogna procedere subito alle gare e che non vale la proroga che abbiamo votato noi, c'è una sentenza del TAR di oggi, che invece dice che i titoli sono validi fino al 2033. Ribadisco che non mi interessa

dei senatori che dovrebbero essere i primi a dire che è la politica che deve decidere quello che succede nel nostro Paese e invece siete lì pronti a giustificare interventi Noi vogliamo che sia la politica a decidere quale futuro debba avere un settore strategico come quello turistico, delle spiagge e delle concessioni balneari, nel nostro Paese. È questo ciò che noi rivendichiamo: non può essere una sentenza del Consiglio di Stato o di un TAR a stabilire cosa bisogna fare in futuro, anche perché se andiamo a vedere nel merito, addirittura c'è l'organo giurisdizionale che stabilisce che la risorsa non è scarsa, quando la Corte di giustizia europea,

dev'essere affidato in modo inequivocabile al legislatore nazionale. È lo Stato italiano - quindi la legge, il Parlamento, il Governo - che deve stabilire se la risorsa è scarsa o no (certo, in accordo con la Commissione europea, che è quello che in questo momento il Governo sta facendo). Allora, alla luce di un'interlocuzione e della fine di un lavoro che si sta facendo con la Commissione europea per stabilire se la risorsa è scarsa o meno sulla base di alcune controdeduzioni che sono state fatte, ossia che il criterio utilizzato è quantitativo e che invece ce ne vorrebbe uno qualitativo, la sentenza di un organo come il Consiglio di Stato non fa altro che indebolire la posizione che il che il Governo e questa maggioranza stanno tenendo nella trattativa con l'Unione europea. Ciò non è ammissibile a prescindere dalle posizioni in campo; è la politica che deve decidere sul tema delle concessioni balneari

si stabilisce poi cosa sarà; non può essere però tutte le volte la sentenza della magistratura, di un organo di giurisdizione, che va in questa direzione. Lo diciamo

che si rispetti il lavoro che è stato fatto. Il tavolo che è stato istituito per stabilire la mappatura e che ha portato al lavoro del Ministero dei trasporti e ad arrivare alla considerazione che la risorsa ora è scarsa è stato previsto in un emendamento che la Lega ha presentato in quest'Aula, che è stato votato;

tema. Pretendiamo però che venga fatta una norma immediata. Come Lega diciamo che su tutti i provvedimenti che arrivano da adesso in poi, noi presenteremo sempre un emendamento che chiarisce una volta per tutte cosa bisogna fare per uscire da questa totale *impasse*. Lo ribadisco: conclusione della mappatura, in accordo con l'Europa, periodo transitorio e poi, quando la risorsa sarà scarsa,

ringrazio per questa opportunità di cui mi avvarrò per pochissimi minuti. La richiesta di intervenire oggi deriva anche dal fatto che noi assistiamo a un susseguirsi di sentenze molto diverse. Giorni fa, il Consiglio di Stato è stato molto severo, ripetendo un orientamento che già conoscevamo. Arriva però oggi la notizia che il TAR di Bari addirittura rimette in vita, secondo la sua decisione, la proroga al 2033 che era stata fatta

da una sentenza del Consiglio di Stato, che diceva che quella legge andava disapplicata. La Cassazione ha poi in qualche modo non dico rimesso in vita, ma caso rivitalizzato tale proposta, affermando che il Consiglio di Stato non poteva fare quella sentenza. Mettiamoci nei panni, comunque la si voglia pensare, di un imprenditore balneare che deve fare degli investimenti, ha avuto una mareggiata quest'inverno e deve ripristinare un'attività; cosa debba fare, quando il Consiglio di Stato disse "per carità, chiudete tutti subito" e la Cassazione dice invece che il Consiglio di Stato non doveva decidere. Il TAR TAR conta meno del Consiglio di Stato, questo lo sappiamo; tuttavia, il TAR di Bari non è che non lo sappia che c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato pochi giorni fa, ma sostiene che la proroga debba avvenire fino al 2033. Ora, cosa deve fare un'impresa balneare di Monopoli? La sentenza

però - voglio che restino agli atti queste considerazioni - in una sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2023, al punto 43 (qui non stiamo facendo discorsi

ha fatto un accertamento e ha stabilito che la risorsa non è scarsa, ma che ci sono spazi per nuove imprese, le quali, se vogliono intraprendere questa attività, lo possono fare; il Consiglio di Stato ha detto che la risorsa invece è scarsa: ma è valido il monitoraggio fatto dal Governo, con la decisione che prese il Governo Conte di prorogare al 2033 le concessioni, o ha ragione

di fare i controlli di sicurezza, ci arresterebbero. Eugenio Scalfari voleva abolire il Consiglio di Stato; non lo hanno ascoltato, quel consiglio non è stato recepito. Non lo faccio mio, però mi chiedo come mai il Consiglio di Stato neghi l'evidenza del monitoraggio, il TAR non ne tenga conto a Bari e l'Europa ("l'ha detto l'Europa") al punto 43 della sentenza che sulla risorsa scarsa il monitoraggio può essere nazionale. E qui mi fermo. Noi tuteliamo delle imprese, che servono al turismo italiano e che devono pagare le concessioni giuste. Non è neanche vero

dal TAR. Forse aveva ragione Scalfari, forse bisogna abolire sia il Consiglio di Stato sia il TAR, ma insomma questo Governo ha aumentato le concessioni e la giustizia amministrativa ha cancellato l'aumento. Serve un po' di ordine, perché un TAR dice una cosa, il Consiglio di Stato ne dice un'altra, l'Europa è severa, ma nella sentenza della Corte di giustizia c'è il punto 43 (studiatevelo). Io credo che tutelare delle imprese in questo caso sia legittimo; è un compito del legislatore, se glielo lasciano fare, e anche del Governo. Quindi rivolgiamo a noi stessi e a tutti un appello a tutelare imprese che creano lavoro e sviluppo. Speriamo che la stagione turistica che si avvicina possa essere vissuta con certezza da chi crea lavoro e accoglie famiglie italiane e turisti stranieri.

nella situazione delle spiagge, la responsabilità è solo vostra. *(Applausi)*. Presidente Romeo, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dalla Costituzione. Bisogna leggerlo tutto l'articolo 1 e non è la sentenza del Consiglio di Stato ad aver dichiarato l'abdicazione del potere del Parlamento. È il diritto dell'Unione europea che ci dice da anni che c'è una regola che si chiama concorrenza che va applicata. Vi abbiamo detto quando c'era il milleproroghe e in occasione della legge di delegazione europea che, se non volevate mettere in difficoltà tutto il settore turistico e balneare, non dovevate continuare con la proroga delle concessioni che sono sotto una procedura di infrazione.

per non mettere in difficoltà la stagione turistica, ma questo lo dovevate fare nel milleproroghe. Non avete sentito quello che le opposizioni vi dicevano, ma non avete sentito neanche quello che il Presidente della Repubblica vi diceva, invitandovi a cautelare di più l'argomento, perché era soggetto a quello che poi era inevitabile, cioè la sentenza del Consiglio di Stato che ora annulla

Bolkestein doveva essere un'opportunità per migliorare la qualità delle nostre offerte turistiche; doveva essere un'opportunità per migliorare i litorali e l'offerta che diamo ai turisti che vengono in Italia; doveva essere un efficientamento di qualità per alzare il livello dell'offerta e della visione turistica del nostro Paese. Invece, per l'ennesima volta e anche oggi in quest'Aula, continuo a sentir parlare di un modo sbagliato di affrontare il tema.

anzi, lo capisco - perché si vuole gettare nel caos per l'ennesima volta il settore balneare. È per una mera strumentalizzazione politica prima delle elezioni. Quello è un settore che invece ha bisogno di certezze e noi continuiamo a trascinarlo avanti con mancate risposte.

diate loro le direttive per fare i bandi. *(Applausi)*. Questo è ciò che va fatto in questo momento. È tutto scritto: gli emendamenti che ha presentato il MoVimento 5 Stelle vi danno per filo e per segno la traccia da seguire.

- quelli presenti in Commissione bilancio, ad esempio - alla discussione in cui abbiamo dovuto affrontare la questione proposta dalla Lega, quando anche la maggioranza aveva difficoltà ad affrontare questo tema, la colpa è tutta vostra, perché io sono preoccupato per la questione degli imprenditori e dei lavoratori. Voi non potete scaricare sugli altri l'incapacità di proporre a tempo debito una soluzione che desse una risposta a quanto poneva

TAR e li mettete in discussione, ma la politica deve rispettare la separazione delle responsabilità, quindi non potete venire a porre questa questione. Voi scaricate sulla giurisdizione l'incapacità di aver affrontato la questione, visto che ci era stata posta. Siete stati incapaci perché,

vista giurisprudenziale, che però non potete mettere in discussione in questo modo. E non venite qui a tirar fuori questo problema, scaricandolo sull'opposizione, quando ce l'avete tutti voi in casa. Quindi, se siete in grado, fate una proposta, ne discutiamo e vediamo quale soluzione trovare,

eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Durnwalder, se intende intervenire. Signor Presidente, mi permetto di ripercorrere brevemente la questione. La richiesta di sequestro del tribunale di Firenze è diretta ad una serie di messaggi scambiati con *e-mail* e *chat* WhatsApp, delle quali viene allegato un elenco, che vedono come interlocutore il senatore Matteo Renzi ed alcuni deputati, relativi ad un periodo temporale ampio, all'incirca dal 2012 al 2019. Tali comunicazioni sono state rinvenute all'interno dei dispositivi informatici sequestrati ad alcuni finanziatori della Fondazione Open, nonché nel corso della perquisizione avvenuta presso lo studio legale del Presidente della stessa Fondazione. Secondo l'impostazione dell'autorità giudiziaria, tale richiesta di sequestro è stata proposta in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, la quale, nel decidere il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della procura di Firenze in relazione al sequestro di alcune conversazioni che vedevano come interlocutore lo stesso senatore, ha chiarito che i messaggi di posta elettronica e WhatsApp, già ricevuti e letti dal destinatario, conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente, hanno natura di corrispondenza fino a quando, per il decorso del tempo, essi abbiano perso il carattere di attualità. Pertanto il tribunale, qualificando come corrispondenza le comunicazioni in premessa, peraltro già estratte dai dispositivi elettronici sequestrati ai terzi, ha chiesto l'autorizzazione del Senato, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Il procedimento penale relativo alla richiesta di sequestro vede il senatore Matteo Renzi imputato, in concorso con altre persone, per il reato di finanziamento illecito di cui agli articoli 7 della legge n. 195 del 1974, 1974, 4 della legge n. 659 del 1981 e 110 e 81 del codice penale. In estrema sintesi, viene contestato al senatore Renzi, quale segretario nazionale del Partito Democratico dal 15 dicembre 2013 al 12 marzo 2018, con esclusione del periodo dal 19 febbraio 2017 al 7 maggio 2017, parlamentare dal 23 marzo 2018 e, secondo l'accusa, gestore effettivo della Fondazione Open, ritenuta dall'autorità procedente di fatto articolazione politica organizzativa del Partito Democratico, di aver ricevuto, in violazione della citata normativa, alcuni contributi di denaro, consegnati da finanziatori alla stessa Fondazione e utilizzati per sostenere l'attività politica negli anni 2014-2018. Il senatore, in concorso con gli altri componenti del consiglio direttivo della Fondazione, avrebbe inoltre ricevuto, sempre in violazione della suddetta normativa, a mezzo dell'interposizione fittizia della Fondazione stessa, contributi in forma indiretta consistenti in beni e servizi acquistati da quest'ultima utilizzando i proventi versati dai finanziatori. Tali fatti sarebbero stati commessi tra il 7 novembre 2014 e l'11 luglio 2018. Secondo l'autorità giudiziaria, le comunicazioni in oggetto apparirebbero pertanto rilevanti al fine di apprezzare le relazioni intercorrenti tra il parlamentare, i consiglieri della Fondazione e i finanziatori stessi della stessa, allo scopo di accertare i fatti contestati. La sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, richiamata dall'autorità giudiziaria, è la decisione con la quale la Consulta ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della stessa procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore senza previa autorizzazione del Senato, in quanto mai richiesta, menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Nella medesima sentenza, la Consulta ha respinto la tesi del tribunale resistente, secondo cui si sarebbe di fronte ad una generica acquisizione di documenti, ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, non rientranti quindi nel novero degli atti dell'articolo 68 della Costituzione, ed ha accolto la tesi del Senato, sulla base della propria giurisprudenza, che ha esteso la tutela costituzionale di cui all'articolo 15 e all'articolo 68 anche ai dati esteriori delle comunicazioni, quelli cioè che consentono di identificare autore, tempo e luogo, ovvero i tabulati telefonici, deducendone che, a maggior ragione, tale tutela deve comprendere il sequestro dei messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario. Tale operazione consente infatti di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle telecomunicazioni, ma anche del loro contenuto, dunque con attitudine intrusiva intenzionalmente maggiore. A supporto di tale conclusione, la Corte ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Pertanto, la Corte costituzionale ha concluso che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione tuteli la corrispondenza dei membri del Parlamento, ivi compresa quella elettronica, anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità in rapporto all'interesse della sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico. Di conseguenza, per tale punto la Corte ha dichiarato che non spettava alla procura di Firenze sequestrare ed acquisire agli atti del procedimento penale la corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp e da messaggi di posta elettronica, annullando il relativo atto di sequestro. La Corte ha anche fornito indicazioni procedurali chiare ai giudici su come eseguire la richiesta di autorizzazione al sequestro sulla base dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Qualora, nell'ambito di un sequestro di dispositivi elettronici di terzi non parlamentari, l'autorità giudiziaria riscontri la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare, deve sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo o dalla relativa copia e chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare, a norma del richiamato articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Nel caso in questione, in realtà, il tribunale di Firenze ha già acquisito il materiale probatorio senza interpellare *ex ante* la Camera di appartenenza del senatore Renzi, avendo quindi già conoscenza del contenuto dei messaggi di testo inviati tramite WhatsApp e posta elettronica. Circostanza anomala e irrispettosa delle prescrizioni della Corte costituzionale, che corrobora le considerazioni in merito alla conclusione raggiunta per il diniego di sequestro. Analizzando infatti le numerose pronunce della Corte di Cassazione che sono intervenute nella medesima vicenda della Fondazione Open, oltre che la stessa sentenza della Consulta sopraindicata, la Giunta è addivenuta all'affermazione della presenza di un *fumus persecutionis* da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti del senatore Renzi, qualificato dal ripetuto e non corretto esercizio del potere di indagine. Si tratta di un *fumus* di contesto specifico e puntuale, reso evidente da diverse pronunce della Corte di cassazione su vicende relative alla Fondazione Open. Si premette che la dottrina e la giurisprudenza parlamentare distinguono tre tipologie di *fumus persecutionis*: il *fumus* di primo grado, inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato, dovuta, ad esempio, ad una inimicizia o ad una avversione personale; il *fumus* di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atta a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus* stesso, ad esempio dalla ripetizione di azioni investigative sul medesimo titolo di reato, tutte terminate con decisioni favorevoli all'indagato; infine, il *fumus* di terzo grado, attinente alle manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. Nel caso della richiesta di sequestro di corrispondenza relativa al senatore Matteo Renzi si ravvisa una tipica figura sintomatica in grado di evidenziare il *fumus* di secondo grado, ovvero la ripetizione di atti di ricerca della prova, specie quando gli stessi risultano illegittimi a seguito del vaglio della Corte di cassazione, che dimostra un'attenzione investigativa eccessiva, caratterizzata da un ripetuto non corretto esercizio del potere di indagine relativo alla Fondazione Open, con la precisazione che la predetta non correttezza emerge, *per tabulas*, dalla lunga serie di decisioni di annullamento pronunciate in tale contesto dalla Corte di cassazione penale. Il rinvio sul punto è alle cinque sentenze citate nella relazione che è già nelle vostre mani. La violazione ripetuta dei principi di diritto affermata nelle sentenze della Corte di cassazione relative alla Fondazione Open costituisce un evidente indice sintomatico di un *fumus persecutionis*, desumibile dall'ostinazione a non uniformarsi alle indicazioni di diritto della suprema Corte. gli elementi evidenziati emerge un quadro sintomatico piuttosto articolato, caratterizzato da un attacco investigativo al senatore Renzi e alla Fondazione Open, con una pluralità di atti investigativi puntualmente annullati dalla Cassazione per una serie di carenze evidenziate con precisazione nelle sentenze richiamate nella relazione sottoposta all'Assemblea. In considerazione di tutte queste motivazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione, a seguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. **Saluto

Signor Presidente, onorevoli colleghi è la terza e, fortunatamente, ultima volta che ho la responsabilità di intervenire sulla vicenda Open. Nel primo caso, nel dicembre 2019, sono intervenuto per avvertire di un pericolo, che era quello del mancato rispetto della separazione dei poteri. è stato per porre il tema di fronte alla Corte costituzionale, nel febbraio del 2022, e oggi per votare. Si chiude, dunque, una vicenda umanamente molto dolorosa e voglio sgombrare il campo da ogni dubbio. Per il processo, qualsiasi cosa voi decidiate, onorevoli senatori, non cambierà niente, perché, al termine della votazione, io depositerò messaggi oggetto della contestazione, anche ove voi votiate, come credo logico e naturale, per respingere l'autorizzazione. E se questo vi sembra un atto di sfida nei confronti dei pm, sappiate che è esattamente così, nel senso che, ritenendo questo processo una farsa senza precedenti, io, una volta che il Parlamento avrà posto la parola fine a questa storia dicendo che non c'è diritto di violare l'articolo 68 della Costituzione, comunque prenderò questi quattro messaggi e WhatsApp e li metterò agli atti. Ciò affinché nessuno possa dire un domani che questo processo finisce per la mancata autorizzazione. Questo processo finisce perché non doveva neanche iniziare, ma è una vicenda che mi vedo io a parte. Non vengo a mettervi in campo le discussioni che riguardano la dinamica processuale; sappiatelo per votare in piena libertà. Ci sono cinque argomenti, li tocco rapidamente. Il primo è che non è della farsa processuale che siamo chiamati a occuparci, ma dello scandalo istituzionale. Ripeto per l'ultima volta: nel settembre 2019 lascio il mio partito per fondare una nuova comunità politica; due mesi dopo 197 finanzieri, alle ore 7,30 del mattino,

responsabili, colpevoli soltanto di aver finanziato in modo trasparente una fondazione che organizzava l'evento politico Leopolda. Questo finanziamento avveniva attraverso dei bonifici bancari; pertanto, ove si fosse voluto prendere la copia del bonifico, si sarebbe potuto limitarsi a chiederla in banca. No, si fanno perquisizioni con 197 finanziari (oggi neanche un'operazione sulla 'ndrangheta ha 197 finanziari), 197 finanziari), che vengono mandati con grande schieramento di forze e tutti i *talk show*, i tg, i *media* per giorni e giorni aprono sul cosiddetto scandalo Open. Contemporaneamente - apro e chiudo una parentesi perché resti agli atti (sono certo che non interesserà la stampa) - in quelle stesse ore, per la prima volta

nel 2022 farà una denuncia e che porterà alla critica di quel cosiddetto metodo Striano. Si sappia - non lo ha scritto nessuno - che la prima volta in cui questa vicenda si verifica in Italia non è sullo scandalo Open, ma è su un accesso abusivo al mio *database,* fatto - ho ragione di credere - casualmente dalle stesse persone implicate nella vicenda Crosetto. Questa storia non è nel procedimento Open; se dico questa cosa è perché so di cosa sto parlando. Si mettono nella stessa identica ora insieme la vicenda Open e una storia che non c'entra niente, che è l'acquisto della mia casa, fatto evidentemente dal sottoscritto e da sua moglie, ma su cui ci sono un accesso abusivo e la pubblicazione di materiale casualmente nello stesso momento. Lo dico perché resti agli atti per il futuro. Nel novembre del 2020 io ho già fatto il mio primo intervento da non indagato. Da quei banchi dico che è uno scandalo l'atteggiamento della procura di Firenze, che vuole disciplinare le forme della politica, per le ragioni che sto per indicarvi. parlo da non indagato, perché sarò indagato soltanto nel novembre del 2020. Un minuto dopo essere indagato, consapevole del mio ruolo di ex Presidente del Consiglio e di membro del Senato della Repubblica, quindi di rappresentante delle istituzioni, mi rivolgo con rispetto al procuratore aggiunto, dottor Luca Turco, titolare dell'inchiesta. Gli scrivo qualcosa del seguente tenore: signor procuratore, come ella sa io sono un parlamentare della Repubblica, vedo dai giornali

a rispettare le procedure della Carta costituzionale, dando da subito la mia disponibilità a votare a favore dell'eventuale richiesta di autorizzazione a prendere il materiale che mi riguarda, perché non ho niente da nascondere, ma siccome sono un parlamentare della Repubblica e l'articolo 68 della Costituzione non è una mia guarentigia, ma è una guarentigia delle istituzioni, del Senato, del Parlamento, prendo carta e penna, metto la firma e dico che lei ha il dovere di rispettare la Costituzione. Accade una cosa incredibile, che se soltanto il Consiglio superiore della magistratura aprisse la pratica disciplinare nei confronti del procuratore che il ministro Nordio ha iniziato, ma che si è persa nella discussione del CSM, sarebbe interessante domandare perché quel procuratore risponde a tutte le istanze che io gli faccio tranne che a questa. Il procuratore, se fosse stato convinto della bontà delle sue azioni, avrebbe potuto dire: caro senatore, o meglio caro indagato, lei non ha alcun titolo per citare l'articolo 68, perché non va bene, io ho diritto di prendere le carte a quel punto si sarebbe chiaramente posto al di là della legge e io dico della Costituzione. Oppure, avrebbe potuto dire: ha ragione, interrompo e apro la procedura chiedendo al Senato della Repubblica l'autorizzazione a prendere il materiale. Questo avrebbe dovuto fare un procuratore della Repubblica che avesse voluto rispettare la legge e la Costituzione, ma non lo fa e non mette per iscritto il diniego alla mia richiesta (perché io sono impeccabile nelle forme e nella sostanza, non scappo dal processo, metto tutto nero su bianco). Se il procuratore della Repubblica Luca Turco avesse seguito la legge e la Costituzione, noi non saremmo arrivati qui oggi, non avremmo dovuto chiedere alla Corte costituzionale di decidere sul conflitto di attribuzione. Avremmo avuto un procedimento corretto. Invece no: la procura di Firenze decide di andare diritto dunque c'è bisogno della sentenza della Corte costituzionale che dice che non è giusto quello che è stato fatto. Ora, questa sentenza della Corte costituzionale - lo ricordo a me stesso per ricordarlo a voi per l'ultima e definitiva volta, amici e colleghi arriva dopo che cinque sentenze della Corte di cassazione hanno detto che il sequestro del materiale da parte dei 197 finanzieri del novembre 2019 non soltanto è illegittimo,

che la Corte di cassazione, non il comitato dei probiviri di Italia Viva, dice ai pm di Firenze: avete preso i telefonini di persone non indagate, con 197 finanzieri tolti dalla strada, dagli uffici o dalla lotta alla criminalità, per andare a capire in modo non consentito se c'è qualcosa sotto agli amici di Renzi. Tu hai dato un contributo alla Leopolda? Benissimo, io vengo a casa tua alle 7 del mattino, ti prendo il telefono, ti perquisisco gli uffici, vado a vedere il tuo telefonino e questa cosa un pm non la può fare e non semplicemente per una ragione di *privacy* sacrosanta, ma perché la legge non permette tutto ciò. Se voi non capite che in questa vicenda non c'è la persona di Matteo Renzi che, vivaddio, se la gode ampiamente per i fatti suoi, ma c'è il vostro futuro

intende stabilire e disciplinare le forme della politica e anche qui c'è un'invasione nei vostri campi.

in modo legittimo, trasparente e regolare da persone fisiche o società a una fondazione. La Fondazione è trasparente, registrata e presenta il proprio bilancio.

senza mancanza di trasparenza. Tutto è legittimo e regolare. Tali denari vanno a una fondazione. Dov'è allora l'elemento per il quale la procura di Firenze interviene? È straordinario. La procura di Firenze decide che quella fondazione non è una fondazione, ma è un partito, o meglio è un'articolazione di partito? la procura di Firenze rivendica agli inquirenti il diritto di disciplinare le forme della politica che la Costituzione, all'articolo 49, ha rimesso non soltanto nella titolarità del Parlamento, ma che il costituente stesso basta aver seguito i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente - fatica a disciplinare stante il grande dibattito culturale e filosofico tra la Democrazia Cristiana *in primis* e il Partito Comunista su come disciplinare un partito politico.

tra l'imprenditore che dà i soldi e la fondazione, decidono che non è una fondazione, ma un partito. Vi rendete conto cosa è questo?

Nella sentenza la Cassazione dice che non ci sono prove che sia un partito. Peraltro il partito ha delle regole democratiche interne che la fondazione si guardava bene dall'avere. Voglio essere molto chiaro. Faceva tutt'altra cosa. Quarto punto. In questo preciso dibattito sarà un caso, ma è impegnato un procuratore della Repubblica e siccome io mi posso permettere il lusso della verità e della mancanza di diplomazia, ho fatto nome e cognome e continuerò a farlo perché io non ho paura Si chiama Luca Turco. Nominato procuratore aggiunto della Repubblica di Firenze dal CSM, il cosiddetto CSM Palamara. Nominato procuratore aggiunto di Firenze, è, del tutto casualmente perché io non voglio parlare di *fumus persecutionis*, ma di coincidenze, lo stesso procuratore che chiede l'arresto di mio padre e di mia madre; lo stesso procuratore che chiede di portare a processo per otto anni mio cognato per un presunto scandalo UNICEF, al termine del quale egli stesso, il procuratore, chiede l'assoluzione, dopo otto anni di gogna mediatica; è lo stesso procuratore che mi indaga per una conferenza all'estero reperibile sul sito di Bloomberg e giudicata inesistente; è lo stesso procuratore che indaga mio padre è lo stesso procuratore che indaga mio padre per un traffico di influenze, che mi tiene ventun mesi per un'accusa di falsa fatturazione. Lo stesso nel giro di pochi anni. Ora sarà un caso, ma mio padre arriva a sessantaquattro anni senza aver avuto alcun problema con la giustizia e, casualmente, nell'anno in cui io divento Presidente del Consiglio, la mia famiglia diventa la famiglia di Bonnie and Clyde e diventa la famiglia verso la quale quel procuratore ha una particolare predilezione. Ho dimenticato un avviso di garanzia a mia sorella; fortunatamente, al momento, ne è rimasta fuori mia nonna

ciò che avviene, secondo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Se vede un reato o un'ipotesi di reato, è giusto che indaghi. Bene, io voglio che questo Parlamento, prima di chiudere, rifletta su quello che è accaduto nel settembre 2022, quando questo procuratore, il dottor Luca Turco, è diventato procuratore facente funzioni di capo alla procura di Firenze. Accade che un immobile, situato in via Maragliano, quartiere 1 di Firenze (non proprio il centro storico, ma nelle immediate vicinanze del centro storico), viene occupato abusivamente. Il Comune di Firenze, la DIGOS e le Forze dell'ordine chiedono alla procura di intervenire per sgomberare. La procura di Firenze, guidata dal dottor Turco, evidentemente impegnata a leggere i ricorsi in Corte costituzionale o in Corte di cassazione, non interviene. Non interviene per settimane e mesi. Quel luogo diventa sempre più un luogo di malaffare e di criminalità. Crescono le richieste di sgombero, ma la procura di Firenze non si occupa di dare una risposta di giustizia ai cittadini che chiedono lo sgombero. Nel maggio 2023 (sono passati otto mesi), un occupante abusivo dell'immobile abusivamente occupato vola dal terzo piano, mentre c'è un regolamento di conti tra le bande che si affrontano dentro l'ex Astor.

Finché il 10 giugno 2023, data tatuata nel cuore di chi ama Firenze (perché Firenze è la città che ha sempre accolto i bambini all'Istituto degli innocenti, dai tempi del Medioevo e del Rinascimento fino a Zeffirelli e agli altri),

è stata rapita o portata via (non sappiamo) arriverà lo sgombero di quell'immobile. Perché vi ho raccontato la storia di Kata, che non ha niente a che vedere con Open? Perché questo è ciò che provano i cittadini che non possono parlare in Parlamento, in tribunale o sui giornali. Vedono il concentrarsi delle attenzioni su una vicenda che non ha niente di sostanziale, decine e decine di finanzieri, centinaia e centinaia di migliaia di euro sprecati in ricorsi e controricorsi, quando chiaramente non c'è niente, e con il Parlamento costretto almeno tre volte a occuparsi di questa vicenda. Però, nel frattempo, una bambina sparisce, un cittadino vola dal terzo piano e non si dà giustizia come si sarebbe dovuto dare. Questo è il punto fondamentale per me. Io non ho problemi da porre oggi alla vostra attenzione. Ho soltanto da domandare a questo Parlamento se intende ricordarsi che c'è una Carta costituzionale, c'è un articolo 68, ma c'è anche e soprattutto un principio di garantismo. Lo dico oggi, in un giorno particolare per il dibattito del Paese. Si è garantisti quando si è garantisti con gli avversari politici, non con gli amici. Quando si è garantisti solo con gli amici, si è ipocriti. Il garantismo si esercita quando si va con gli avversari. Questo è un passaggio difficile, perché a noi il garantismo non ce l'avete dato, neanche voi che oggi fate sfoggio di questo. Non ci avete fatto professione di fede garantista quando ci sono stati gli scandali (o presunti tali) legati alle banche, legati a Open e legati alle vicende della famiglia. Noi siamo orgogliosi di essere stati garantisti con voi, anche quando voi non siete stati garantisti con noi. Ma quello che è certo è che o siamo garantisti o la politica avrà perso la propria dignità, perché la dignità della politica - ed è la ragione con la quale - ed è la ragione con la quale concludo il mio appello - è quella che porta a dire che questa vicenda ha distrutto la mia *privacy*, persino il conto corrente, ha messo a dura prova la vita della famiglia, perché potete immaginare cosa voglia dire spiegare a dieci nipotini che i nonni sono stati arrestati (e poi liberati dopo dieci giorni). Il TG1 che apre con l'immagine della stanza dell'interrogatorio, in violazione di tutte le leggi e di tutti i codici di deontologia professionale. Ha violentato i miei finanziatori ha danneggiato il mio partito. Noi abbiamo perso nel giro di una settimana la metà delle stime dei sondaggi, immediatamente: il 19. Ovvio, in televisione non si parlava più di politica, si doveva spiegare come avevo comprato la casa o perché avevo fatto un acquisto con la carta di credito. Questa vicenda, però, non ha fatto venire meno, almeno in me, la voglia di continuare a combattere perché questo sia

e si cerchi di attuarlo. Non so se questo è uno dei miei ultimi interventi in questo Senato, ma mi piace pensare che sia l'ultimo su Open. Dopo tre interventi, non auguro a nessuno di passare quello che abbiamo passato noi, ma dico a chi ce l'ha fatto passare che noi siamo sempre i soliti: sorridenti, tenaci e gagliardi. Quello che è certo, però, è che se questa cosa, anziché andare su delle spalle che possono reggere il peso

Comunque votiate, sappiate che non si sta discutendo di me, ma ricordatevi che si sta discutendo della dignità del Parlamento della Repubblica, della dignità del Senato della Repubblica, della dignità delle nostre istituzioni. Buon lavoro a tutti voi.

Signor Presidente, come è stato anticipato dal relatore, la Giunta ha compiuto un'attenta disamina sulla vicenda che il senatore Renzi poc'anzi stava ricordando in maniera anche chiaramente emozionata, riguardandolo personalmente e riguardando gli affetti più cari che una persona si trova attorno, soprattutto nel momento nel quale si sa di aver subito probabilmente un grave torto

relazione che poc'anzi il relatore ci ha specificato andando poi a concludere proponendo il respingimento della richiesta di sequestro in questione - che questa disamina ha certamente tutta la possibile nostra preoccupazione per gli aspetti che la magistratura si trova quotidianamente a dover dirimere e regolamentare. Siamo poc'anzi usciti da una discussione che riguardava l'intervento sull'economia, sull'aspetto collegato alla disciplina delle gare della Bolkestein e la questione dei balneari, che guarda caso vede dei magistrati dirimere o tentare di farlo, perché si è dimostrato come ci siano addirittura anche tra Corti della stessa natura amministrativa diverse visioni del problema. Abbiamo visto come la magistratura - lo ricordava il senatore Renzi - possa intervenire a gamba tesa su vicende che hanno a che fare anche con la legittimazione diretta da parte del popolo dei rappresentanti che devono andare andare ad amministrare la cosa pubblica, e quindi anche sulle libertà che vengono conseguentemente limitate, a fronte di esercizio dell'attività giurisdizionale. Naturalmente

nella Carta costituzionale. Sono delle limitazioni poste dalla Carta costituzionale, a ben vedere, sull'azione invasiva e intrusiva, che può essere naturalmente anche legittima, della magistratura. Ma probabilmente il Costituente, dopo le note vicende in materia politica e bellica che vedevano l'Italia uscire da una guerra civile, aveva ben visto la necessità di porre un freno a quelle azioni che potevano anche rivolgersi nei confronti di soggetti eletti nelle sedi parlamentari e che per ciò solo lo avevano probabilmente stimolato

l'organo di appartenenza dell'eletto per rappresentare le ragioni di un esercizio giurisdizionale a carico di un parlamentare. Non siamo qui, ovviamente, a difendere la categoria, non lo vogliamo certo fare, ma nel momento in cui addirittura la Corte costituzionale, che va ad interpretare queste norme, riconosce e qualifica dei contenuti

all'attenzione del magistrato come possibile materiale dal quale estrarre dei convincimenti che non sono corroborati fino a quel punto, ma che si presume lo possano diventare in ragione delle conversazioni scambiate tra soggetti, peraltro estranei all'indagine, ebbene in quel momento anche la Corte costituzionale si sente si sente motivata nel dare la propria lettura dei fatti. Lo fa naturalmente anche limitando il soggetto inquirente nella possibile qualifica della natura della fondazione nei rapporti con i partiti politici. Lì si apre una vicenda ancora più dettagliata, perché si intende specificare che manca del tutto la motivazione per la quale si ritiene che quel soggetto giuridico, facente funzioni di un ente come la fondazione, possa essere

che vengono sviluppate all'interno della nota sede della Leopolda. Ebbene, è evidente non può non trovarsi d'accordo con la serie continuativa di pronunciamenti della Cassazione, che in quel momento vanno a costituire quella "plausibilità" - così la definisce il relatore che rende evidente trovarsi di fronte ad una situazione veramente paradossale, in quanto l'insistenza dell'organo inquirente e poi naturalmente anche le tesi del tribunale del riesame, che tendono a confermare quella lettura inquisitoria, vanno a costituire anche quella verosimiglianza che noi, membri della Giunta, dobbiamo utilizzare per rendere estrinseci gli elementi del *fumus persecutionis*. non posso che trovarmi d'accordo quando il relatore, dando una compiuta esposizione dei famosi tre gradi del *fumus persecutionis*, che vengono appunto individuati attraverso una in quanto funzione primaria - attività persecutoria del magistrato, quando appunto si chiama *fumus* di primo grado, una modalità di azione promossa al di fuori delle ragioni di un'azione persecutoria e di un'azione promossa in sede giudiziaria non motivata - e quindi siamo di fronte a un *fumus* di secondo grado - e infine un *fumus* di terzo grado quando siamo davanti alla manifesta infondatezza dell'azione.

la stessa ragione dell'azione senza altri punti indiziari e qualificano quella persecutorietà dell'azione giudiziaria che noi siamo chiamati a identificare identificare e a rendere motivo della decisione di diniego della Giunta. È ovvio che tutta questa storia

*ad nutum* a poter chiudere una prima archiviazione istruttoria o addirittura una soluzione per scarsa rilevanza, mancando lo *strepitus fori*.

esca con una assoluzione con formula piena da una vicenda giudiziaria assurda che, guarda caso, riguarda un'altra Open. Ebbene, ricordando anche persone che non sono più tra noi come Giovanni Paolo Bernini, che per tanti anni ha fatto della sua vicenda giudiziaria un motivo di lotta che lo ha portato che lo ha portato probabilmente nel dolore anche a morire prematuramente, io ritengo che quella che ha definito la Giunta del Senato sia una vicenda dalla quale prendere assolutamente spunto per il futuro.

Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la Giunta, da massimo consesso paragiurisdizionale a cui è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione e alla valutazione delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, oltre a quello di esaminare le domande di autorizzazione a procedere e di quelle relative ai reati ministeriali, si è trasformata - ahimè e sottolineo ahimè nell'organismo politico per eccellenza. Oramai ci troviamo di fronte ad un organo che, in base alla mera convenienza politica e non allo studio delle carte, istruisce e consegna all'Assemblea il verdetto da votare. La maggioranza ci sta mostrando che tutto può essere strumentalizzato. Tutto può essere o bianco o nero o grigio, a seconda della convenienza politica del momento. Non fa eccezione, purtroppo, la materia del contendere. Per la prima volta in questa legislatura - e non lo dico perché vi sia stata una convenienza politica, ma sarà sicuramente frutto del caso - la relazione conclusiva della Giunta si basa quasi esclusivamente su pronunce della magistratura. Fino ad ora i lavori in Giunta sono stati mossi da interpretazioni giuridico-politiche volte a rivedere le valutazioni dell'organo giudiziario al fine di escludere l'applicabilità delle richieste provenienti da quest'ultimo. Adesso avviene il contrario. Siccome nel caso in specie le sentenze della Cassazione potevano essere utilizzate come elemento a favore della deliberazione volta al diniego dell'autorizzazione a procedere, esse sono state quasi integralmente riproposte nella relazione. Tale questione, utile ai fini del caso di specie, ha suscitato però forti preoccupazioni in Giunta, tant'è che - come da resoconto sommario - sia il senatore Scalfarotto che la senatrice Spelgatti hanno sollevato preoccupazioni in merito al fatto che la Giunta, per i futuri casi, non dovrà essere vincolata da sentenze della Cassazione per quel che concerne il *fumus persecutionis*. Sarebbe come voler dire: in questo caso seguiamo la Cassazione, perché le sue decisioni possono essere prese come pezze di appoggio per avanzare la proposta di diniego all'autorizzazione a procedere; ma non fossilizziamoci troppo su queste ultime, poiché poiché ce ne potrebbero essere alcune che, invece, siano tali da giustificare un'eventuale decisione a favore della concessione dell'autorizzazione. Insomma, gli elementi vanno analizzati caso per caso, ma a seconda della mera convenienza politica, a tutto danno della certezza del diritto. Diciamo che, relativamente a questo modo di intendere le regole, l'attuale maggioranza non teme confronti. Un ultimo esempio di equilibrismo politico istituzionale si è avuto in Commissione affari costituzionali della Camera, laddove era in corso di votazione il provvedimento sull'autonomia differenziata o meglio lo "spacca Italia". Il Presidente di Commissione, non curante del fatto che si fosse raggiunta la maggioranza per l'approvazione di un emendamento a prima firma di un componente del MoVimento 5 Stelle, ha interrotto le votazioni e riconvocato la Commissione per il giorno successivo. Bel modo di legiferare: piegate la realtà a vostro piacimento. Altro esempio: tutti sanno che lo sviluppo dell'Italia necessita del Mezzogiorno. Una crescita equilibrata e di qualità del Sud assicura un grande beneficio all'intero territorio nazionale. siete più preoccupati del voto di scambio tra premierato e autonomia differenziata che delle sorti dell'Italia. Complimenti: state piegando le istituzioni a vostro comodo e per di più a Costituzione invariata. Figuriamoci cosa accadrà con il premierato. A proposito di premierato, colgo la palla al balzo, perché qui in Aula abbiamo il fautore dell'ultima riforma costituzionale, colui il quale avrebbe dovuto abbandonare la politica se il *referendum* del 2016 non fosse andato in porto. Non pensiate di raggiungere un risultato diverso qualora doveste avere l'ardire di approvare in duplice lettura la vostra riforma costituzionale. Torniamo a noi. La relazione conclusiva del relatore offre una valutazione che il Gruppo che ho l'onore di rappresentare non condivide. Richiamando una ripartizione in tre tipologie di gradi del *fumus persecutionis*, si apprezza lo sforzo del relatore nell'aver ripreso una dottrina minoritaria che si è palesata in un paio di occasioni nel 2015. Il cosiddetto *fumus persecutionis* di secondo grado, quello che motiverebbe la presente deliberazione, si manifesta quando le modalità particolari dell'azione promosse dai magistrati siano atte a far trapelare, da elementi oggettivi, la parvenza della persecuzione: così dal resoconto sommario della seduta della Giunta del 18 febbraio 2016. dov'è il *fumus* nei confronti del senatore Renzi? Ci sono state per caso modalità particolari delle azioni promosse da magistrati che facciano trapelare la parvenza della persecuzione? quello che si evince dalla lettura delle carte non si direbbe. Sul punto, esprimo valutazioni diverse da quelle del relatore. La prima Facendo seguito alla sentenza della Consulta, che ha equiparato *chat* ed *e-mail* alla corrispondenza, il gup del tribunale di Firenze ha richiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione al sequestro in relazione all'ipotesi di reato di finanziamento illecito. Non avrebbe potuto fare tale richiesta *ex ante*, come invece erroneamente si ipotizza nella relazione conclusiva, in quanto, prima della sentenza della Corte costituzionale, la n. 170 del 2023, la giurisprudenza qualificava gli atti oggetto della richiesta come documenti, quindi, estranei rispetto al concetto di corrispondenza, quest'ultima sì rientrante nelle guarentigie di cui all'articolo 68 della Costituzione. La seconda valutazione: il *fumus* deve essere circoscritto al soggetto verso il quale la deliberazione ha gli effetti. Nella relazione conclusiva si qualifica la presunta persecuzione in ragione dei provvedimenti emessi dalla Suprema corte, che in alcuni casi ha cassato, con o senza rinvio, le diverse deliberazioni del tribunale del riesame in merito all'applicabilità del sequestro di dispositivi elettronici. Ebbene, anche in questo caso, dove è il *fumus* nei confronti del senatore Renzi? Che c'entra con il *fumus* il fatto che vi siano stati dei provvedimenti della Cassazione che hanno annullato le pronunce del tribunale del riesame in relazione a soggetti terzi rispetto al senatore Renzi? Il sequestro può essere considerato come onnivoro o invasivo nei confronti dei privati finanziatori - mi rifaccio a quanto riferito alle pagine 8 e 9 del documento conclusivo del relatore - e invece come indispensabile per il senatore Renzi, al fine di appurare se le *chat* e le *e-mail* contenute nel dispositivo siano rilevanti nell'apprezzamento delle relazioni intercorrenti tra il parlamentare, i consiglieri della fondazione e i finanziatori della stessa, e nel valutare le funzioni e le finalità delle donazioni in ragione del fatto di escludere eventuali collegamenti col sostegno della sua attività politica esclusiva e dei parlamentari a lui vicini. Siamo anche stupiti del fatto che il senatore Renzi abbia annunciato comunque che depositerà in giudizio il citato materiale, a prescindere dalle valutazioni del Senato. Siamo stupiti, ma fino a un certo punto. Del resto, anche lo stesso senatore ha annunciato, quando è stato audito in Giunta, la prossima prescrizione. È giusto? Attraverso lei, signora Presidente, auguriamo al senatore Renzi di essere eletto alle consultazioni europee, ma gli ricordiamo che a Bruxelles vigono sensibilità e regole severe in materia di conflitto di interessi. Per queste ragioni, non reputando sussistere gli elementi oggettivi atti a sostenere la tesi di *fumus persecutionis,* esprimo il voto contrario alla relazione conclusiva del relatore.

ben delineato l'ambito di descrizione di quello che si intende per corrispondenza. È chiaro che, da quando è stata scritta la Costituzione ad oggi, sono intervenute delle modifiche

i nuovi strumenti come ricadenti appieno nell'ambito della corrispondenza. Se non fosse stato così, saremmo arrivati a intendere il contenuto della corrispondenza veramente in uno strettissimo ambito, ovvero quello della corrispondenza cartacea, della lettera,

e dalla riconoscibilità del soggetto interessato dal provvedimento. È chiaro che nel conflitto di attribuzione il Senato difende le prerogative non del singolo senatore, ma dell'istituzione parlamentare

dunque il conflitto di attribuzione e richiesto che il provvedimento di sequestro dovesse passare attraverso la Camera di appartenenza del senatore, arriviamo così a discutere del tema.

Vi sono vari livelli per considerare il *fumus*, che sono stati prima anche ampiamente illustrati dal senatore Durnwalder al relatore, che tra l'altro ringrazio anche per il lavoro che ha fatto su un tema che richiede un particolare equilibrio

non può non essere considerato una persecuzione nel momento in cui ogni provvedimento che viene fatto e sistematicamente annullato dalla Cassazione poi venga ripresentato e venga di nuovo sanzionato dalla Corte di cassazione

dall'amicizia o dall'inimicizia. È chiaro che poi possono essere coinvolte le singole storie che delle volte denunciano delle realtà che sono dei fatti. Il problema in sé non è la condanna: se interviene la condanna, è chiaro che va rispettata; una condanna non va commentata e una sentenza va semplicemente eseguita. Il problema è quando i processi nascono sulle indagini e chi ricopre cariche pubbliche, chi ha versi, anche l'onere di rappresentare i propri cittadini e di lavorare nel mondo della politica, è particolarmente esposto. Queste macchine che iniziano con delle indagini hanno spesso portato alla distruzione di carriere, di persone e famiglie, magari poi per arrivare al nulla. Non si sta dicendo di non fare i processi: si sta dicendo di fare i processi con la tutela delle garanzie. È quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto con molti provvedimenti della Commissione giustizia proprio nell'ultimo anno e penso che questo sia un percorso che dobbiamo costantemente continuare con equilibrio.

Presidente, cercherò di evitare di ripetere tante cose che già sono state dette. In particolare è stato ricordato da tutti, anche dalla collega Stefani e dal senatore Renzi, che quella odierna è la seconda volta che quest'Aula esamina un documento che riguarda l'inchiesta della Fondazione Open e il senatore Renzi. Quest'Aula si era espressa già nella scorsa legislatura quando sollevò il conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Firenze per il sequestro delle *chat* del senatore Renzi. Quel conflitto di attribuzione portò a quella famosa sentenza che è stata illustrata testé dalla senatrice Stefani, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto che le *chat* e le *e-mail* non sono meri documenti, ma sono corrispondenza e quindi, come tali, devono essere sottoposte alle guarentigie previste dall'articolo 68

prima di questa sentenza della Corte costituzionale si riteneva pacificamente che le *e-mail* e le *chat*, anche quelle di WhatsApp, fossero mera documentazione e quindi sequestrabili liberamente e non sottoposte ai limiti del sequestro della corrispondenza. l'argomento che viene utilizzato per cui il tribunale di Firenze si sarebbe comportato illegittimamente sequestrando direttamente le *chat* e le *e-mail* è infondato perché il tribunale di Firenze agì sulla base di una giurisprudenza costante, che poi è stata innovata dalla Corte costituzionale con sentenza apprezzabile, con la quale è stato invece riconosciuto che quel tipo di documentazione è in realtà assimilabile a corrispondenza e quindi, come tale, come tale, deve avere anche i limiti della corrispondenza e quindi essere sottoposto anche ai limiti previsti all'articolo 68 della Costituzione. Per questo siamo tornati a occuparci della questione per verificare

*fumus persecutionis*. Ora sul punto, a prescindere dal fatto che - come ha detto il senatore Renzi - la scelta che assumeremo noi sul piano pratico, che riguarda il processo in sé, è irrilevante, irrilevante, perché - come ha dichiarato ripetutamente il senatore Renzi - egli depositerà quelle *chat* ed *e-mail* comunque agli atti - quindi dal punto di vista processuale la nostra decisione è ininfluente - è molto importante invece

ben cinque sentenze della Corte di cassazione, che hanno riguardato esattamente sequestri disposti dalla procura di Firenze nell'ambito dell'indagine sulla Fondazione Open. Quelle sentenze si sono ripetute, talune anche costrette a farlo sullo stesso sequestro, perché per due volte la Corte di cassazione ha stabilito che il sequestro fatto dalla procura di Firenze di Firenze nell'ambito dell'inchiesta era illegittimo e ha invitato la procura a uniformarsi ai principi di diritto che stabiliva la Corte di cassazione. E per due volte la procura ha ignorato i rilievi della Corte di cassazione, la quale alla fine, con la terza sentenza riguardante il medesimo sequestro, è stata costretta a cassare senza rinvio il provvedimento di sequestro, continuando a ritenere che si trattasse di un sequestro illegittimo. Questo per dire quanto la Corte è stata costretta a intervenire. È importante ricordare i rilievi che ha fatto la Corte di cassazione nell'annullare ripetutamente i provvedimenti di sequestro della procura di Firenze. È già stato detto - ma penso sia opportuno ribadirlo - che la Corte di cassazione ha anzitutto ritenuto che mancasse il cosiddetto *fumus commissi delicti*: ha cioè ritenuto che il tribunale non abbia mai provato adeguatamente la tesi che sta alla base dell'inchiesta, cioè che la Fondazione Open fosse uno schermo fittizio dietro il quale si nascondeva un'articolazione del Partito Democratico o fosse essa stessa direttamente un'articolazione del Partito Democratico. La Corte di cassazione ha detto che questa tesi non è in alcun modo suffragata da elementi indiziari, con i quali il tribunale doveva confrontarsi prima di emettere un provvedimento di sequestro. Per ben cinque volte, nelle sentenze che si sono ripetute (da ultimo nella sentenza del 2022), la Corte di cassazione ha detto che non c'era il *fumus commissi delicti* e quindi ha fatto crollare la tesi sulla quale si fonda l'inchiesta della procura di Firenze. Ma non solo. Come è stato ricordato, la Corte di cassazione ha ripetutamente stigmatizzato le modalità

di sequestri a carattere esplorativo, cosa non consentita. I sequestri si fanno per acquisire elementi probatori e indiziari definiti e predefiniti; non si fanno a strascico per eventualmente valutare, se dentro la pesca a strascico, si trova qualche elemento indiziario. Quindi, non si fa un sequestro a carattere esplorativo e sproporzionato, cioè non proporzionato al sacrificio dei diritti di *privacy* e di libertà delle persone alle quali sono stati sequestrati le *chat*, le *e-mail* e i cellulari, rispetto alla necessità di accertare il reato. Ha parlato anche ripetutamente di un sequestro onnivoro - stiamo parlando appunto di un sequestro eccessivo

tanto vero che, alla fine, la Corte di cassazione è stata costretta ad annullare il sequestro senza neanche rinviare al tribunale per riesaminare il provvedimento. A noi pare che tutti questi elementi concorrano nel ritenere fondata la valutazione che ha fatto il relatore nel documento che ha proposto alla Giunta e ora viene proposto all'Aula. In termini all'Aula. In termini di plausibilità - noi non dobbiamo accertare che ci sia una persecuzione in atto, ma dobbiamo semplicemente accertare se dagli elementi che ci sono stati forniti è plausibile ritenere che forniti è plausibile ritenere che ci sia un *fumus persecutionis* - a noi pare che gli elementi siano abbastanza limpidi nel supportare la nostra valutazione, che è di consenso rispetto alla proposta del relatore. Pertanto voteremo a favore della proposta.

intervengo a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per illustrare la serie di ragioni per le quali la vicenda giudiziaria che afferisce al senatore Renzi riveste indubbiamente una valenza particolare in termini regolamentari, in termini di diritto parlamentare, in termini di giurisprudenza costituzionale, ma anche in termini strettamente politici. Riveste una particolare rilevanza proprio in funzione della necessità di tutela delle prerogative irrinunciabili e, in quanto tali, indisponibili connesse alle funzioni parlamentari e, quindi, nella disponibilità e nella tutela dell'Assemblea e del singolo parlamentare. La vicenda che occupa oggi l'Assemblea e che la impegna alla responsabilità del voto attiene non alla persona del senatore Renzi quanto piuttosto al tema estremamente delicato e dirimente della necessità di bilanciamento di due interessi contrapposti, entrambi costituzionalmente tutelati: da un lato, il diritto-dovere di svolgere investigazioni giudiziarie in ambito penale e, quindi, la necessità di tutelare il vincolo reale, il sequestro degli eventuali elementi di prova; dall'altro lato, però, però, la valutazione della necessità di comprimere il diritto, la libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare. Questo naturalmente prescinde del tutto dalla persona fisica del diretto interessato, dal suo ruolo politico, dalla sua notorietà giudiziaria, dalla sua collocazione ideologica, dalla sua presa di posizione politica. Dobbiamo tutti partire da un presupposto necessario per il quale l'articolo 68 della Costituzione, anche in tema di autorizzazione preventiva al sequestro di qualunque forma di corrispondenza, anche informatica, di un parlamentare della Repubblica, offre delle guarentigie, insieme alla legge n. 140 del 2003, che sono a tutela primaria della sovranità e dell'indipendenza dell'Assemblea legislativa rispetto a potenziali aggressioni da qualunque altro organo o potere dello Stato, e soltanto successivamente e strumentalmente a tutela della persona che in quel momento rivesta la pubblica funzione. Questo comporta che la nostra valutazione oggi in Aula debba sfumare dalla tutela della posizione del senatore Renzi, arrivando a valutare invece i rischi costanti dell'esistenza del *fumus persecutionis*. Mi riferisco alla possibile aggressione alla sfera dell'indipendenza dell'organo legislativo da parte del potere dell'autorità giudiziaria. È questo il tema indifferibile che dobbiamo porci quest'oggi. E, rispetto al tema del *fumus persecutionis,* noi abbiamo un'evidenza talmente incidente e massiva da aver comportato, da un lato, l'intervento della Corte costituzionale (è stata ricordata la sentenza n. 170 del 2023, che ha stabilito una volta e per tutte che qualunque forma di comunicazione afferisca alla posizione di un parlamentare vada salvaguardata con l'autorizzazione preventiva della Camera alla quale appartiene) un numero impressionante di pronunce di merito da parte del tribunale del riesame e della libertà. Vi sono state inoltre ben sei, se non sette pronunce di legittimità da parte della suprema Corte di cassazione, che ha espresso parole lapidarie, che sono la mortificazione per un determinato modo di svolgere la funzione giudiziaria, quando si parla di uso «esplorativo» dei mezzi di ricerca della prova; quando si giunge a ritenere che l'attività di una procura della Repubblica abbia assunto caratteri invasivi o onnivori, e quindi privi di qualunque controllo; quando è possibile che perfino il relatore alla Giunta delle elezioni e delle immunità, di ben altro schieramento politico, abbia potuto argomentare - certo in termini di plausibilità e di verosimiglianza di un quadro sintomatico di un attacco investigativo alle garanzie di un parlamentare della Repubblica. Allora, dinanzi a questo scenario, di assoluta inquietudine per un'Assemblea parlamentare, dinanzi alla quale massima dovrebbe essere l'attenzione dell'Assemblea sovrana, soltanto una fortissima dose di irresponsabilità, unita certo a un'altrettanta forte dose di cinismo, può permettere di derubricare quanto sta accadendo a una sorta di epitaffio funerario nei confronti del senatore Renzi: «*Sic transit gloria mundi*». Noi in questo momento dobbiamo essere liberi da questa forma di irresponsabilità e di cinismo, perché il cinismo è proprio e soltanto di chi conosce il prezzo di ogni cosa e non conosce il valore di nulla. Noi, invece, da destra ancora oggi confermiamo di avere forte il senso delle istituzioni; di avere l'apprezzamento e il faro della Costituzione; di apprezzare fino in fondo la forza delle leggi e di avere il coraggio della lealtà verso l'avversario politico, anche quando questo non sarebbe conveniente. Abbiamo il senso della responsabilità che, nel nostro caso, è l'etica della responsabilità, che deve sempre accompagnarsi all'orgoglio e al culto dell'appartenenza. Per noi sarebbe stato molto semplice e comodo partecipare al rito dello sciacallaggio e contribuire ad azzannare alla gola il mostro di Firenze. Avremmo potuto tranquillamente infierire, forti della copertura e dell'alibi di una così invasiva procedura giudiziaria. Ma noi abbiamo un'altra *forma mentis*, un'altra statura, un'altra forma di correttezza nei confronti dell'avversario politico. Allora, nonostante i numeri ce lo consentissero, sia in Giunta che oggi in Aula, noi rifiutiamo la tesi dell'abdicazione rispetto al ruolo del quale siamo consapevoli protagonisti. Avremmo anche potuto abbandonare il senatore Renzi al suo destino. «Faccian le bestie fiesolane strame di lor medesime». Ma noi non abbiamo inteso farlo, perché rivendichiamo fino in fondo la dignità del ruolo parlamentare la forza, la costanza, la pienezza del ruolo parlamentare. E si badi: i temi sollevati con l'inchiesta giudiziaria alla base di questa attività così invasiva sarebbero stati degni di maggiori approfondimenti: i rapporti del Partito Democratico con la Fondazione Open ritenuti opachi; l'equivoco del finanziamento alla Fondazione Open; i rapporti del senatore Renzi con i responsabili della Fondazione, la sistematica messa a disposizione da parte della Fondazione e a favore di parlamentari del Partito Democratico di carte di credito e di carte bancomat come come risultanti dall'inchiesta; il famoso volo ricco di suggestioni, pagato per il senatore Renzi verso Washington; 135.000 euro, pagati non si sa a che titolo dalla dalla Fondazione Open a favore di un soggetto che non risultava il titolare del potere decisionale. Ma soprattutto, dietro una possibile attività di accertamento giudiziario, c'era il tema, delicatissimo, del finanziamento ai partiti e se quindi la Fondazione potesse essere considerata un'articolazione del Partito Democratico attraverso la quale aggirare il divieto di finanziamento pubblico previsto dalla legge. Ma se questi sono gli argomenti, noi ci siamo dovuti inchiodare alla responsabilità quando abbiamo preso atto della legge costituzionale, dell'articolo 15 della Costituzione, dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E, quindi, in questo senso, noi, Presidente, voteremo voteremo a favore della proposta del relatore di diniego dell'autorizzazione per un ordine di fattori ben evidente, e uso le parole del senatore Renzi: noi sappiamo distinguere la giustizia dal giustizialismo, le garanzie dalla gogna. Noi abbiamo il coraggio e la visione romantica di affrontare e sconfiggere il nemico sul piano politico. Per dirla come Indro Montanelli: noi siamo ancorati a una visione romantica della vita e della politica, per cui continuiamo a preferire, se necessario, "le zanne delle belve alla bava degli sciacalli".

per il quale è pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi un procedimento penale per diffamazione dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo alla relatrice, senatrice Stefani, se intende intervenire.

un prefigurato reato di diffamazione a carico del senatore Matteo Renzi a seguito di una querela presentata dal dottor Francesco Basentini, magistrato della procura di Potenza, ex direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avrebbe effettuato, a riguardo della citata procura, nell'ambito della cosiddetta indagine Tempa Rossa, nonché sulla nomina dello stesso dottor Basentini a capo del DAP da parte del Ministro della giustizia. Si evince che questa querela sia stata sporta a seguito di alcune dichiarazioni fatte dal senatore Renzi durante una trasmissione televisiva del 29 maggio 2022.

durante questa trasmissione televisiva. Il magistrato, a seguito dell'istanza, ha due vie da scegliere: una è di decidere e di considerare che sussista la prerogativa parlamentare; oppure, nel caso in cui ritenga che questa non vi sia o abbia dubbi riguardo alla medesima, può deferire la decisione alla Camera di appartenenza, in questo caso il Senato. Vi è un ulteriore modulo procedurale, che è il caso in cui lo stesso senatore possa attivare *motu proprio* e promuovere egli stesso la decisione della Giunta. Nel caso di specie, nonostante le sue ripetute istanze, il senatore Renzi, non avendo avuto una risposta, ha ritenuto di avvalersi della procedura speciale, quindi di attivare e di promuovere direttamente la decisione della Giunta. Sul piano sostanziale, dobbiamo ancora ricordare, com'è già noto a quest'Assemblea, che, come costante giurisprudenza della Corte costituzionale, affinché possa sussistere l'insindacabilità, occorre che vi sia innanzitutto un nesso funzionale

Abbiamo potuto verificare che, sempre nel caso, il senatore Renzi era intervenuto, durante la seduta del Senato del 20 maggio 2020, proprio sulle mozioni di sfiducia nei confronti dell'allora ministro della giustizia Bonafede.

Nella seduta dell'Assemblea, quindi, aveva più volte ricordato l'attività che era stata svolta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, soprattutto rispetto alle scarcerazioni durante il periodo Covid-19.

Riteniamo, poi, che sussista anche il requisito temporale, in quanto fra la dichiarazione esterna, resa nel corso della trasmissione televisiva, e quella resa all'interno di quest'Aula vi sia un lasso di temporale piuttosto ridotto. Abbiamo svolto ovviamente in Giunta la discussione e l'analisi della della questione in esame. La Giunta ha quindi deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi il procedimento penale per diffamazione davanti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza concerna opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che pertanto viga nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Signor Presidente, non solo è interessante che quest'oggi ci occupiamo di due casi che riguardano lo stesso nostro collega, il senatore Renzi; ma in realtà credo sia interessante la di quest'oggi perché ci siamo occupati di due aspetti diversi dell'articolo 68 della Costituzione. Nel primo caso, abbiamo dovuto decidere sulla possibilità di sequestrare la corrispondenza di un parlamentare; adesso, ci occupiamo invece dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Devo dire che questo dell'insindacabilità è un caso più semplice, nel senso che anche la giurisprudenza

da un parlamentare all'esterno del Parlamento corrispondono in via funzionale a ciò che egli ha detto *intra moenia*, quindi all'interno dell'istituzione, quelle opinioni non possono essere soggette a un giudizio penale. Quello che affrontiamo oggi, che riguarda la causa intentata dal dottor Basentini nei confronti del senatore Renzi, come diceva bene la collega Stefani, è proprio il caso di scuola, perché Renzi ha espresso delle opinioni circa l'operato in particolare del DAP allora diretto dal dottor Basentini e quelle dichiarazioni erano state molto simili a quelle espresse non soltanto in un dibattito parlamentare, ma addirittura in un dibattito sulla fiducia al ministro della giustizia Bonafede e quindi per la Giunta la decisione è stata abbastanza semplice.

Anche in questo caso, nonostante l'interessato fosse un membro del Parlamento e avesse fatto rilevare di essere un senatore, quindi di dover godere delle guarentigie

parlamentare nel suo complesso, singolarmente il giudice non ha tenuto conto dell'istanza presentata dall'indagato, cioè dal senatore Renzi, il quale pertanto ha dovuto utilizzare una norma della legge ordinaria che dà esecuzione all'articolo 68, quindi è soltanto per questo che siamo arrivati a decidere in Giunta sulla questione. Sollevo questo punto perché nel dibattito precedente ho trovato ho trovato molto interessanti alcuni rilievi che sono stati fatti, tali per cui si è data la colpa alla Giunta di essere larga di manica. Ora, essere larghi di manica e allargare eccessivamente il significato e la portata della norma costituzionale è probabilmente un comportamento che non va tenuto, ma devo dire che ancor peggio

Non c'è il *fumus persecutionis*, se un parlamentare viene attaccato con provvedimenti giudiziari che per cinque volte la Corte di cassazione ritiene illegittimi? Sottolineo che la Corte di cassazione non è soltanto fatta da magistrati, ma è la più alta istanza giurisdizionale del Paese, quindi ci riferiamo non soltanto a dei magistrati, ma a dei signori magistrati. Non c'è *fumus persecutionis* perché

in questo caso nemmeno l'insindacabilità, come non c'è mai stata in nessun caso. Oggi abbiamo avuto l'ulteriore ipotesi di un ex senatore

Noi dobbiamo metterci un po' d'accordo: o la Costituzione italiana è la più bella del mondo sempre o non lo è. Quando la Costituzione italiana decide di proteggere la funzione parlamentare e la libertà dei parlamentari di esercitare la loro attività di rappresentanti del popolo, tale norma esprime la medesima bellezza che noi vediamo promanare dall'intera Costituzione. Diventa allora molto sospetto

chiunque, qualsiasi imputato, sia innocente fino a sentenza passata in giudicato, avere una sentenza di condanna di primo grado sulle spalle non è certamente piacevole e non lo è in particolare per chi esercita un'attività pubblica politica come un parlamentare o un ex parlamentare.

degli aspetti ideologici e di parte e di ricordarci che tra le nostre responsabilità c'è anche quella di preservare la funzione parlamentare e di passarla alle prossime legislature così come l'abbiamo ricevuta da quelle precedenti, di non abdicare mai al prestigio del Parlamento, di non rinunciare mai alla sua libertà e di non accettare mai invasioni di campo da altri poteri dello Stato, che queste Camere rispettano sacralmente. Infatti noi davanti all'autogoverno e all'autonomia della magistratura ovviamente ovviamente ci fermiamo, però, così come noi ci fermiamo davanti a quelli, dobbiamo pretendere - non per noi, ma per l'istituzione che rappresentiamo, che è la massima istituzione di di rappresentanza popolare - che le prerogative del Parlamento siano sacralmente rispettate. Per tali ragioni, voteremo a favore della relazione della collega Stefani.

e dunque il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle sulla richiesta di insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Renzi in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza. Cercherò di illustrare le motivazioni. Signor Presidente, a discapito di quello che hanno detto alcuni colleghi, abbiamo provato a spiegare le nostre motivazioni, ma a quanto pare non abbiamo convinto i membri della Giunta. Non ci sono riuscita. È un dato di fatto, siamo stati l'unico Gruppo parlamentare che ha votato contro.

quelle risatine, perché siamo gli unici che, come sempre, ribadiscono il no, continuamente e convintamente solo per principio. Ci ridono sopra

che il Gruppo che io rappresento non è il partito che dice no per principio. Proverò a spiegare in dieci minuti che non siamo i seguaci del no a tutto, ma che siamo un

Andiamo ai fatti e ai lavori della Giunta. Stavolta voglio entrare proprio in maniera quasi banale e diretta diretta sui fatti e sui lavori che abbiamo affrontato in Giunta. Il pubblico ministero di Potenza Giuseppe Borriello ha disposto la citazione a giudizio per il senatore Matteo Renzi, per la diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'ex capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, in riferimento all'inchiesta cosiddetta Tempa Rossa condotta proprio dal magistrato nel 2016. Quali sono state le parole che hanno portato Basentini a fare questa denuncia? Sono state le parole proferite da Matteo Renzi, intervistato in una trasmissione condotta da Massimo Giletti, "Non è l'Arena", il 22 maggio 2022 (specifico le date), proprio in merito alla vicenda delle dimissioni di Francesco Basentini. Leggo testualmente le parole usate da Renzi: «Ora che Basentini non è più a capo del DAP, qualcuno dovrebbe farsi delle domande sulla famosa inchiesta Tempa Rossa. Il suo merito, agli occhi della maggioranza di allora, fu proprio quell'inchiesta fuffa. Ci fu un enorme dispiegamento di forze, vennero pubblicate intercettazioni sulla vita privata delle persone, la bravissima ministra Guidi fu costretta a dimettersi, eppure l'indagine non portò a nullaۛ». Continua il senatore Renzi (testuali parole): «L'obiettivo non era fare un processo, Basentini ha organizzato, indagato partendo da una presunta ipotesi di reato, è stato protagonista di un buco nell'acqua e, come premio, è andato al DAP». Parliamo ora di questa inchiesta, Tempa Rossa. In quell'inchiesta fu indagato Gianluca Gemelli, all'epoca compagno della ministra dello sviluppo economico del Governo Renzi, Federica Guidi, che proprio in seguito agli sviluppi di quell'inchiesta si dimise. Per l'accusa, Gemelli aveva commesso il reato di traffico di influenze illecite, perché, approfittando della convivenza con la Ministra, avrebbe ottenuto promesse, requisiti e qualifiche necessari a partecipare alla gara per i lavori dell'impianto estrattivo di Tempa Rossa. Secondo le intercettazioni telefoniche, Gemelli sarebbe stato rassicurato dall'ex Ministra in merito all'inserimento di un emendamento, che poi fu presentato nel 2014, con

le opere connesse alle attività estrattive di gas e petrolio erano di interesse nazionale, prevedeva uno snellimento delle procedure e dell'*iter* per il via libera alle attività industriali, una specie di meccanismo

Nel decreto viene specificato che, dopo l'avviso di conclusione delle indagini parlamentari, Renzi ha richiesto di rendere interrogatorio, che però in due occasioni, il 6 ottobre e il 13 ottobre 2023 (perché il processo è ancora in corso), non si è svolto per l'assenza dello stesso Renzi, che una volta ha presentato un legittimo impedimento, la seconda volta invece senza giustificarlo, né documentarlo. Il 13 novembre 2023, data indicata dallo stesso Renzi per presentarsi all'interrogatorio, che egli stesso aveva indicato come richiesta di rinvio, non si presenta e contestualmente rinuncia all'interrogatorio e riporta le memorie difensive depositate dal suo avvocato di fiducia.

un collegamento e un nesso funzionale tra le parole usate nella trasmissione televisiva

con il suo intervento in Aula del 20 maggio 2020, in virtù della mozione di sfiducia nei confronti dell'allora ministro della giustizia Bonafede, che facevano riferimento alla questione della scelta del vertice del DAP e alla gestione delle carceri al tempo del Covid.

al Ministro, il senatore Renzi si limitava a denunciare una certa superficialità nella gestione del Covid nelle carceri, alludendo a un suo suggerimento - inascoltato - al Ministro della giustizia per la nomina del DAP. Nel citato intervento, dunque, non veniva non veniva in nessun modo fatto riferimento all'inchiesta Tempa Rossa condotta dal magistrato nel 2016, né tanto meno si ventilava un'ipotesi di complotti giudiziari addebitati allo stesso nel maggio del 2022. Queste sono le motivazioni per cui abbiamo votato contro la relazione proposta. *(Applausi)*. In nessun modo c'è coincidenza contenutistica, né tantomeno connessione funzionale, tra le dichiarazioni rese in Assemblea e quelle rese nella trasmissione televisiva. Non ci sono neanche altri atti *intra moenia* di Renzi e, in generale, azioni politiche dell'ex *Premier* che rimandino vagamente alla vicenda Tempa Rossa o al ruolo avuto

la posizione politica del *premier* Renzi fu del tutto opposta. Basta fare una ricerca su Internet e si trovano le parole utilizzate dal *premier* Renzi nei confronti dell'allora ministra Guidi.

un errore. Non c'è niente di illecito ma ha fatto un errore e ne va preso atto. In Italia adesso chi sbaglia va a casa». Io dico: magari|! *(Applausi)*. Mi accingo a concludere, Presidente, e voglio

Rilevo che la Commissione che deve giudicare sull'applicazione dell'articolo 68 ha da tempo adottato una linea di condotta sulla quale è opportuno fare una riflessione sincera.

salvando così i parlamentari dall'eventuale processo: l'immunità non è mai stata negata a nessun parlamentare di qualsiasi partito; sembra quasi che ci sia un tacito accordo secondo il quale tutti salvano tutti, perché oggi io salvo te e domani tu salvi me. *(Applausi)*. È una logica che è ben distante dalla natura stessa dell'articolo 68 della Costituzione, il cui scopo è - o, meglio, doveva essere -quello di impedire che la libertà dei parlamentari venga limitata dalle autorità giudiziarie. Era quindi un articolo...

Sono veramente perplessa e colpita dall'atteggiamento tenuto in Aula anche dalla collega che mi ha preceduto. Vorrei soltanto ricordare, per suo tramite, Signor Presidente, alla collega e a tutto il MoVimento 5 Stelle che quello che noi dobbiamo fare in Giunta è attenerci strettamente alla Costituzione. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, tutela la libertà la libertà delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni: è una garanzia costituzionale. La Costituzione non la si può invocare quando si vuole e dimenticare in altre occasioni. Noi dobbiamo limitare l'esame, quando siamo in Giunta, soltanto a due fattori per applicare la prerogativa dell'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione: se c'è il nesso funzionale tra le opinioni rese *extra moenia*, quindi fuori dal Parlamento, rispetto a quello che è stato detto in Parlamento e se c'è una un legame temporale rispetto alle dichiarazioni. Il caso che oggi trattiamo, quello del senatore Renzi, rispecchia esattamente questi due criteri, per tutte le motivazioni che sono state dette prima. Noi

non è fatto per coprire qualcuno o per garantire qualcuno, ma per garantire la libertà di espressione dei parlamentari che sono stati eletti dai cittadini. È quindi il sistema democratico che viene tutelato in questa maniera. La spiegazione del motivo per cui certe posizioni vengono tenute in Giunta o di quello che è stato detto oggi l'ha fatta la stessa collega precedentemente, nel momento in cui ha detto espressamente: dico a chi ascolta. Questi sono discorsi che non hanno nulla a che vedere con l'ambito giuridico che deve essere applicato nel caso concreto e quindi con la Costituzione, le sentenze giurisprudenziali e tutti i precedenti che stabiliscono a che cosa dobbiamo attenerci,

in estrema sintesi, l'articolo 68, a saperlo leggere e comprendere, dice che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nel corso delle funzioni parlamentari. Per comprenderlo, basta semplicemente avere un minimo di senso delle istituzioni, non essere succubi delle pronunce e delle richieste dell'autorità giudiziaria e non essere adusi al "servo encomio" ed al "codardo oltraggio"; poiché *intelligenti pauca*, esprimo il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

per il quale è pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi un procedimento penale per diffamazione dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la

Signor Presidente, onorevoli senatori, la settimana scorsa è venuto a mancare Stefano Stefani, figura storica della Lega e uomo politico di primissimo piano. Senatore per due legislature, tre volte deputato, Presidente della Commissione affari esteri della Camera, Stefani ha ricoperto importanti ruoli di Governo come Sottosegretario all'ambiente e come Sottosegretario alle attività produttive in due Governi Berlusconi. Imprenditore di successo, presidente federale della Lega Nord, Stefani è stato un punto di riferimento importantissimo per tutti i militanti e i dirigenti della Lega, soprattutto per noi veneti. Protagonista di mille battaglie, uomo di lotta e di Governo, sempre in prima fila nella battaglia per la libertà e l'autonomia del Nord e del Veneto, Stefani è stato un esempio di passione politica, di dedizione e di generosità. A nome del Gruppo Lega, esprimo alla famiglia la nostra vicinanza e il nostro profondo cordoglio. Addio presidente Stefani, grande veneto, grande vicentino, grande leghista.

Signora Presidente, in quest'Aula abbiamo avuto modo diverse volte di discutere della nostra sanità e dei problemi del sistema sanitario regionale. Spesso dalle opposizioni si attacca la maggioranza, dicendo che hanno intenzione di privatizzare la nostra sanità e, in tutta risposta, sentiamo grandi proclami di la volontà di salvare il nostro sistema sanitario e di tutelare e valorizzare il nostro personale sanitario. questa maggioranza, tramite il suo candidato Presidente e Governatore della Regione Piemonte, sta calando la maschera, perché è di ieri l'annuncio dell'attuale e forse futuro - ahinoi presidente del Piemonte Cirio, che ha dichiarato a Torino la nascita di un pronto soccorso gestito da privati. E via: dopo che l'aveva annunciato l'assessore alla sanità Icardi, smentito dallo stesso Cirio, oggi è lo stesso Cirio a dichiarare di voler consegnare i pronto soccorso del Piemonte alla sanità privata. Questo è un primo passo. Ci sarà un un bando nei prossimi mesi, entro ottobre, e chissà che cosa seguirà. Ecco che cade quindi la vostra maschera e dichiarate innocentemente, strizzando l'occhio in campagna elettorale alla sanità privata, che della salute dei cittadini piemontesi, ma anche italiani, non ve ne frega